Sono anni che si aspetta un intervento, dopo che era stata fatta la legge del 1994, che aveva sicuramente delle buone intenzioni, ma che nei fatti non ha avuto i risultati sperati. Questa è una legge quadro che ha delle misure concrete per la montagna. Da bergamasca, anche se sono donna di pianura, questa legge per noi è molto importante. Ringrazio innanzitutto un altro bergamasco come me, il ministro Calderoli, per il grande lavoro fatto

questa legge affronta tantissime tematiche e quindi sono tanti i Ministeri coinvolti nella definizione del testo e degli emendamenti. È stato fatto un lavoro certosino e gli emendamenti sono stati valutati uno a uno, sia per la Commissione che per l'Aula, che per l'Aula, che fossero della maggioranza o dell'opposizione. Credetemi che c'è stato il massimo impegno per far sì che il testo, che già comunque aveva un ottimo impianto con le sue misure fondamentali, fosse ulteriormente migliorato. Il testo

armi e delle misure concrete che possano servire ai territori montani per svilupparsi da un punto di vista economico al fine ridurre i divari territoriali. Non è una legge assistenzialista, ma è una legge che dà

poco conto della fatica che si fa a vivere e a lavorare in montagna, perché è tutto più complicato, e non solo da un punto di vista climatico, ma anche per gli spostamenti, le infrastrutture e quant'altro. Proprio per questo bisogna prestare una grande attenzione alla tutela dei servizi, partendo innanzitutto dall'istruzione e dalla sanità, incentivando lo sviluppo economico e sostenendo il tessuto socioeconomico. Una grande attenzione è stata data alle imprese giovani,

Con la precisa definizione di montagna si vanno a ridurre gli sprechi e si cercherà di applicare le misure al meglio, prevedendo un continuo monitoraggio per capire anche quanto occuperanno a livello economico tutti gli interventi

legge. Ricordiamo però che - come precisato nel corso dell'esame in Commissione - una delle finalità fondamentali è agevolare l'accesso ai servizi pubblici essenziali, in particolare sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connessione e mobilità; promuovere in maniera sostenibile l'agricoltura e la gestione forestale, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo; valorizzare il patrimonio culturale e montano

estendendo l'attività di promozione anche allo sviluppo sostenibile. L'articolo 2 reca norme per la definizione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani in base al parametro altimetrico della pendenza per la creazione di uno o più elenchi dei Comuni montani, perché i Comuni montani non hanno tutti le stesse necessità. Un ulteriore decreto andrà a individuare i Comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione e l'elenco dei Comuni montani beneficiari. Sempre grazie all'esame in Commissione è stata introdotta la delega al Governo a riordinare la normativa vigente in materia di agevolazioni, anche di natura fiscale, in favore dei Comuni montani. dei Comuni montani. L'articolo 3 reca la definizione della strategia nazionale per la montagna italiana, che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Ancora in Commissione, è stato previsto un parere da parte delle Commissioni competenti per materia. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento degli interventi da parte del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, dal 2025 sono ripartiti questi fondi tra Regioni, enti locali e poi poi ci sono le misure di competenza statale. Il Dipartimento per gli affari regionali, in base all'articolo 5, avrà il compito del monitoraggio dell'attuazione e dell'impatto delle disposizioni, e si prevede la presentazione alle Camere di una relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della strategia entro il 28 febbraio di ciascun anno. All'articolo 6 si introducono due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari che lavorano nei Comuni montani, a cui viene attribuito un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera nelle procedure concorsuali; è prevista una valorizzazione nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l'assunzione di incarichi; sono previsti un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di 2.500 euro per coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna o vi effettuano il servizio di medico di base - un altro tema fondamentale - o acquistano con accensione di finanziamento in base agli stessi criteri. In Commissione è stato aggiunto un riconoscimento per i Comuni che presentano delle minoranze linguistiche con un aumento degli incentivi a favore di questi territori. È stato previsto in Commissione uno speciale emolumento per il personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale nei Comuni montani, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta. Si introduce, con l'articolo 7, la definizione di scuole di montagna per assicurare l'autonomia del personale docente dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e il servizio scolastico nelle scuole di montagna. Importantissima novità introdotta dalla Commissione è stata l'eliminazione dell'attuale limitazione territoriale, per cui la possibilità di derogare al numero minimo di alunni per classe - questa è una cosa importantissima - è ammessa nelle istituzioni scolastiche ed educative del primo e del secondo ciclo di istruzione, caratterizzate dalla presenza di alunni con fragilità negli apprendimenti; quindi, si riconosce tale possibilità di deroga anche con riferimento ai nuovi percorsi ordinamentali e percorsi sperimentali della scuola secondaria di secondo grado. Viene dato un punteggio aggiuntivo per le graduatorie provinciali di supplenza per chi ha prestato servizio nelle scuole di montagna, si riconosce un credito d'imposta a favore di coloro che prestano servizio in scuola di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo o acquistano un immobile nei Comuni di montagna, caso il credito d'imposta viene aumentato per i Comuni in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche. Sempre in Commissione, all'articolo 8 è stato introdotto un emendamento che consente al Ministero della giustizia di provvedere alla copertura delle piante organiche dei tribunali siti nelle zone di montagna disagiate con una carenza di organico pari almeno al 30 L'articolo 9, così come modificato dall'esame in Commissione, prevede che le università e le istituzioni AFAM aventi sede nei Comuni montani possono stipulare accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca per promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per la montagna. Le università possono attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza. Poi ci sono altre novità previste dalla Commissione, come il fatto che le università possono promuovere un programma di partenariato per l'innovazione con gli operatori privati, e l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei Comuni montani. Sempre in Commissione, all'articolo 10 si garantisce la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali previste nei contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e si individua, quali strumenti attraverso cui assicurare lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, la copertura della rete Internet in banda ultra larga e il sostegno alla digitalizzazione. L'articolo 11, come modificato dall'esame in Commissione, reca disposizioni sull'adozione di linee guida per individuare, recuperare, utilizzare e valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani. L'articolo 12, sulla disciplina degli ecosistemi montani, riconosce le zone montane come zone florofaunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana. L'articolo 13, come modificato dalla Commissione, prevede la possibilità di destinare una quota del Fondo a interventi di carattere straordinario, anche in coerenza con le misure previste dal decreto siccità, per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità di risorse idriche. L'articolo 14, modificato in Commissione, modifica il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, inserendo la definizione dei cantieri temporanei forestali e l'utilizzazione boschiva. L'articolo 15, introdotto in Commissione, definisce le nozioni di albero monumentale e di boschi monumentali, con le modalità previste per la tutela. L'articolo 16, modificato in Commissione, riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani. Il credito d'imposta nei casi in cui gli investimenti vengano fatti nei Comuni non superiori a 5.000 abitanti è aumentato. davvero importante sulla manutenzione dei territori: sempre l'articolo 16 consente ai Comuni montani e alle forme associative montane l'affidamento diretto dei lavori di sistemazione e di manutenzione del territorio, di gestione forestale, di difesa dall'avversità atmosferiche e dagli e dagli incentivi boschivi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Abbiamo la definizione dei rifugi di montagna e la definizione di percorso escursionistico tanto attesa dai territori, con disposizioni in merito alle attività escursionistiche. Sempre introdotto dalla Commissione, abbiamo un credito d'imposta previsto per le piccole imprese e le microimprese che esercitano la propria attività nei Comuni montani i cui titolari non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero le società e le cooperative i cui soci per più del 50 per cento non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età; ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per più del 50 per cento da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno d'età. L'articolo 22, modificato in Commissione, prevede di agevolare lo svolgimento del lavoro agile nei piccoli Comuni montani e il ripopolamento degli stessi e riconosce uno sgravio contributivo per il datore di lavoro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato che non abbia compiuto il quarantunesimo anno d'età e che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità agile nei Comuni sotto i 5.000 abitanti. Si è introdotto all'articolo 23 un credito d'imposta nel caso di mutuo contratto da un contribuente che non abbia compiuto il anno di età per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia di un immobile da destinare ad abitazione principale. Un altro punto fondamentale è stato inserito in Commissione all'articolo 24, in Commissione all'articolo 24, per agevolare la natalità e contrastare lo spopolamento. È previsto nei Comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti un incentivo per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di uno dei predetti Comuni, dopo l'entrata in vigore della legge, entro il limite di 5 milioni di euro annui, con un contributo *una tantum* il cui importo sarà poi determinato con decreto del Ministro per la famiglia.

di due anni ha varato due importantissimi provvedimenti, attesi da tempo: la legge quadro sull'autonomia per realizzare questa grande riforma e il

Si tratta sostanzialmente di disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane e l'attuazione dell'articolo 44 della Costituzione.

«La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane». Il provvedimento ribadisce che la crescita economica e sociale delle zone montane costituisce un obiettivo di interesse nazionale

intende altresì limitare gli squilibri economici e favorire il ripopolamento. Questo è un grande tema che sta attraversando il dibattito politico degli ultimi decenni. Abbiamo assistito, purtroppo, a un abbandono di molti territori e Comuni di montagna,

la propria residenza) possa vedere nella montagna stessa una grande opportunità di crescita lavorativa e avere anche una vita migliore sotto molti punti di vista, più a contatto con la natura, in ambienti sicuramente migliori rispetto a certi agglomerati urbani. Gli interventi che vara questo provvedimento sono, ad esempio, quelli relativi alla sanità e alla scuola nel tentativo di incentivare i professionisti del comparto scuola e del comparto sanità a esercitare la professione in quelle zone. Quindi, è rivolto anche a incentivare questo meccanismo che permetta ai residenti in montagna di avere servizi essenziali adeguati. L'articolo 2, poi, affronta un grande tema, che è quello della classificazione dei Comuni montani. Da uno studio fatto dall'Unione nazionale Comuni, comunità riportato nella relazione illustrativa, si evince che il territorio montano comprende attualmente 3.524 Comuni totalmente montani e 652 parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 e per un territorio che si evidenzia montano addirittura del Quindi, è evidente che le attuali classificazioni rappresentano un'Italia per metà montana.

sono adeguate se vanno ad aiutare quei Comuni che sono effettivamente montani, per i quali lo stanziamento o meno di quelle risorse comporta effettivamente dei vantaggi o l'ininfluenza delle risorse che vengono stanziate. Credo quindi che vadano utilizzate con maggiore efficacia per i Comuni effettivamente montani mi auguro che l'attività successiva permetta di centrare questo obiettivo, che è fondamentale. È interessante anche l'emendamento che è stato approvato, che assegna una delega al Governo per integrare e riordinare la normativa vigente

abbiamo bisogno esclusivamente di rendere servizi adeguati a chi vive in montagna e magari lavora in città da pendolare, ma abbiamo bisogno anche di favorire che quegli insediamenti economici che esistono ancora oggi in montagna, non necessariamente solo nel campo dell'agricoltura e dell'allevamento, che pure sono fondamentali e importanti e da salvaguardare, abbiano adeguata possibilità di sopravvivere.

che noi riteniamo molto importante, che ha eliminato l'attuale limitazione territoriale per la deroga al numero minimo di alunni per classe, e questo è un grande tema che ha riguardato spesso i Comuni montani. Purtroppo, il calo delle nascite ha fatto sì che alcune classi non avessero il numero sufficiente per sopravvivere, addirittura interi plessi scolastici. Attraverso questa deroga si dà la possibilità ai bambini che nascono e crescono in montagna di poter frequentare la scuola nei propri territori e non doversi spostare magari a lunghe distanze. È evidente che questa è una delle cause principali che potrebbe provocare lo spostamento di intere famiglie dalla montagna in territori dove i servizi scolastici sono più adeguati. Era una deroga attesa da tempo e finalmente in questo provvedimento è stata inserita ed è stata approvata con il contributo del del Parlamento e del Senato della Repubblica. Ci sono poi norme che riguardano non solo la vita quotidiana dei cittadini, ma ma anche la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, la tutela degli ecosistemi montani in una visione molto ampia all'interno del provvedimento. poi una norma, che è frutto di un emendamento presentato dal nostro capogruppo Romeo, che è stata approvata ed è relativa all'articolo 24, che ha inserito gli incentivi per la natalità nei

non è mai sufficiente qualsiasi stanziamento adottato - ma è importante che esista questa norma all'interno della legge, perché dà la possibilità in futuro, qualora gli effetti siano positivi, di poterla incrementare più agevolmente. definitiva, questa legge quadro ha un obiettivo fondamentale, ossia tutelare chi vive e lavora in montagna: chi vive, perché abbia servizi adeguati; chi lavora, perché non fugga da quei territori. Non tutta la montagna può vivere esclusivamente di turismo; ci sono territori fortunati che hanno in questa attività una risorsa fondamentale che fa essere quelle zone montane ricche e prosperose, con redditi molto alti, ma ci sono anche zone montane che vivono di sussistenza, di agricoltura e di allevamento. Ci auguriamo che questo provvedimento tuteli anche quelle realtà, che sono poi la parte preponderante del nostro Paese. signor Presidente. Mi dispiace che non si sia potuto toccare il tema della reintroduzione dei lupi in montagna, che ha creato gravi danni a molti allevatori. Esiste un problema di convivenza, poiché i branchi sono aumentati a dismisura dopo la loro reintroduzione. Ci sono normative europee che permetterebbero in deroga del numero dei lupi, ma l'Italia non le ha ancora recepite. Il Gruppo Lega ha presentato una proposta di legge per adeguarsi alla normativa europea sia alla Camera che al Senato; era iniziato l'*iter* alla Camera, ma è bloccato perché mancano i pareri del Ministero dell'ambiente. Ci auguriamo che finalmente questi pareri arrivino e si vada avanti nell'*iter*, che è fondamentale per permettere a un'attività come quella dell'allevamento di coesistere e permanere in montagna, visto che negli ultimi anni abbiamo avuto una grande riduzione di tali attività e la chiusura di molte malghe, e non credo sia nell'interesse di nessuno. Un plauso va

Signor Presidente, saluto innanzitutto i colleghi presenti e il Governo. Sono ormai decenni che assistiamo al fenomeno dello spopolamento delle aree montane e rurali, sempre più lasciate sole dalle istituzioni a vario livello. Da questa disattenzione sono derivate carenze di infrastrutture; fragilità geologica per scarsa manutenzione e irrazionale consumo del suolo; sanità di prossimità e smantellamento; fuga dei medici verso territori che offrono maggiori prospettive economiche, e non solo: dispersione scolastica e dispersione professionale. Ciò si è tradotto in disuguaglianze, isolamenti, divisioni sociali, povertà. Il disegno di legge in esame contiene sicuramente buoni principi e intenti assolutamente condivisibili, ma ne rinvia l'attuazione a successive iniziative legislative e governative. Oggi parlano in maniera più chiara i contenuti della bozza della nuova legge di bilancio, che dettano una chiara linea di austerità. Il Governo Meloni, infatti, intende penalizzare Regioni e Comuni di oltre 4 miliardi nei prossimi tre anni, di cui 1,6 miliardi solo l'anno prossimo, con gli investimenti agli enti locali che dal 2029 subiranno importanti riduzioni. Sostanzialmente, ancora una volta ci si fa belli e interessati, elencando una serie di buoni propositi, però poi al di fuori di qui ci si prepara a una serie di tagli che non favoriranno assolutamente queste buone intenzioni. Anzi, sono state approvate proposte emendative che lo stesso MoVimento 5 Stelle aveva presentato, tra cui quelle sulle agevolazioni fiscali per l'acquisto di immobili nei Comuni montani a favore di medici e operatori sanitari in generale, forme premiali per i medici che esercitano nei Comuni montani, la possibilità di creare classi scolastiche in deroga al numero minimo di alunni per le scuole in montagna. Occorre, però, evidenziare che le cifre di finanziamento indicate saranno assolutamente e decisamente insufficienti, se consideriamo i corposi tagli dal prossimo anno che ho appena menzionato. A ciò aggiungiamo che si sta facendo poco per supportare le Regioni nella tutela delle fonti idriche e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Sono attualissimi attualissimi gli eventi calamitosi, di cui si parla tanto in questi giorni. Questo è grave, ci preoccupa, ma non è la sola preoccupazione. C'è infatti un altro dato che ci ricorda come il sistema delle comunità montane sia stato smontato; un sistema che comunque assicurava servizi associati tra Comuni, investimenti investimenti per la protezione, per lo sviluppo socioeconomico dei territori. Inoltre, negli ultimi due decenni sono stati rivisti anche i criteri per la definizione dei Comuni montani e si sono realizzate categorie come quella delle aree interne. Sono mutamenti che stanno provocando ulteriore confusione, ulteriore frammentazione delle varie aree del nostro Paese. Precisiamo ancora che questo provvedimento è un passo importante, ma dovrà essere confermato da successive iniziative, al fine di ottenere un miglior coordinamento con le istituzioni territoriali. A tale proposito, la previsione di un tavolo tecnico per l'attuazione di quanto contenuto in questo provvedimento, composto da soli rappresentanti governativi, senza includere, senza contemplare la partecipazione delle Regioni e degli enti locali, dimostra ancora una volta la poca sensibilità che si ha nei confronti delle istanze territoriali, l'assenza di unità e partecipazione tra i vari livelli istituzionali. Inoltre, noi siamo convinti della necessità di un sistema di perequazione negli ambiti territoriali che vada oltre il contesto esclusivamente comunale. Parliamo di una logica sovracomunale e per questo abbiamo proposto proposto un emendamento che avrebbe consentito di estendere alle associazioni dei Comuni l'affidamento dei lavori di sistemazione e mantenimento del territorio montano. Ancora, riteniamo inidoneo e fonte di ulteriori disuguaglianze e di ulteriore frammentazione basare i finanziamenti ai territori solo sui livelli di pendenza e di altitudine e non su aree omogenee, discriminando così i Comuni montani e non montani che presentano comunque le stesse caratteristiche morfologiche e demografiche, considerata anche la presenza di tanti Comuni con la stessa altitudine, ma in aree economicamente e morfologicamente differenti e stanti le medesime necessità di migliaia e migliaia di Comuni, nonostante altitudini differenti. Tale scenario si complica ulteriormente per aver previsto l'esclusione della categoria dei Comuni parzialmente montani dalla possibilità di utilizzare il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Noi abbiamo presentato emendamenti che miravano a ridurre le disuguaglianze tra i Comuni; proposte attente ai territori rurali interessati dalla transizione industriale, che scontano gravi svantaggi, tipici delle zone montane, a causa della difficoltà di adeguamento dei processi produttivi. emendamenti che individuavano i Comuni delle zone montane utilizzando non soltanto il criterio altimetrico, ma anche quello geomorfologico, al fine di includere anche quei territori situati, ad esempio, nel fondovalle, in collina, alle pendici delle montagne. Emendamenti, ancora, che sopprimevano il limite dei 5.000 abitanti, al fine di trattare in egual modo Comuni che condividono le stesse problematiche, pur con una popolazione e con una popolosità magari lievemente differente. Concludo ricordando che stiamo per votare un disegno di legge che ha lo scopo di aiutare ecosistemi ricchi di tradizioni, di arti, di professioni, dalle radici antiche e nobili, ricchi di fonti energetiche primarie (parlo di acqua, legno, vento), con basso inquinamento, beni archeologici e paesaggistici, una biodiversità di pregio mondiale. Occorre pertanto fare una riflessione più ampia, a nostro avviso. Con il tempo si è diffusa la cultura della valorizzazione delle sole mete di eccellenza, riconosciute magari da UNESCO o da altre istituzioni internazionali altrettanto importanti. È la tendenza a mettere al centro il turismo e politiche urbanistiche orientate principalmente a favorire e a sviluppare le strutture ricettive nelle località turistiche maggiormente gettonate. Tuttavia, al di fuori di questo contesto e di queste reti esiste altro - ne stiamo parlando oggi - appunto le aree rurali e montane, che spesso vengono trattate quasi come un peso, come una zavorra improduttiva. Siamo perciò convinti che questo atto sia sicuramente importante. È necessario adottare - lo ribadiamo - misure volte a valorizzare queste aree e considerare la montagna non solo per il turismo, ad esempio scommettendo sulla filiera del legno e su pratiche di allevamento innovativo che rispettino gli animali e l'ecosistema e realizzino prodotti di alta qualità. È necessario investire sull'importanza dello scarso consumo del suolo come un valore aggiunto e sul lavoro creativo ad elevata innovazione tecnologica. Questo disegno di legge si riduce però a un mero manifesto, ricco sicuramente di buone intenzioni. Ci chiediamo come si coniughino queste finalità, sicuramente nobili, con la scelta del Governo di definanziare ad esempio il fondo per le piccole opere comunali, di ridurre i contributi per gli investimenti in rigenerazione urbana, di tagliare il fondo per i progetti di messa in sicurezza degli edifici pubblici, senza dimenticare i cambiamenti che innescherà necessariamente l'autonomia differenziata e la decisione scellerata - lo ribadisco anche in questa in questa sede - di bandire la coltivazione della canapa industriale, ad oggi tra le attività produttive maggiormente in espansione. Questi esempi dimostrano quanto il Governo Meloni alla fine non sia così favorevole allo sviluppo delle aree montane, perché delibera e legifera in maniera contraria o comunque non utilizzando gli strumenti che potrebbe utilizzare per favorire veramente e concretamente le aree di cui stiamo discutendo oggi. Sostanzialmente si continua a raccontarla bene. Ci raccontiamo sempre una bella storiella (e noi auspichiamo ovviamente che trovi concretezza); però, di fatto, oggi siamo ancora davanti a una bellissima storiella.

la sua sensibilità verso i territori e la sua sensibilità verso i temi che vogliono vedere l'Italia crescere. *(Applausi)*. Credo che il disegno di legge sulla montagna vada proprio in questa direzione. Mi spiace sentir dire dalla collega che mi ha preceduto che sono solo favolette. Ministro, io sono una donna di montagna, provengo da quei territori e questo disegno di legge l'ho letto; c'è tutto quello che serve per dare risposte concrete alla montagna. Lei ha preso tutte le risorse, le normative che c'erano sono state raggruppate in questo disegno di legge proprio per dare le risposte necessarie ai territori e soprattutto a un fenomeno che spesso è sulla bocca di tanti (ma rimane solo sulla bocca), quello dello spopolamento della montagna. Sulla montagna c'è una doppia visione. Una visione è ideologica ed è quella delle persone che vedono la montagna come la cartolina, come la pista da sci, come il territorio dove fare le passeggiate. Ma la montagna non è solo questo. Oddio, la valle da dove provengo io offre questo e - come è stato detto da chi mi ha preceduto - ci sono due tipi di montagna: la montagna in cui si è sviluppata l'economia turistica e che ha avuto modo di crescere e di offrire opportunità di lavoro e la montagna che vive basandosi sull'economia dei paesi che sotto la mantengono. Ma non è questo quello che noi vogliamo. Io mi ricordo, basata anche su questa ideologia ai tempi della pandemia, quando tutte le strutture alberghiere sono state chiuse in inverno, che la reazione di tanti è stata: è solo una sciata. Questo racchiude come venga vista la montagna. Come ha reagito il popolo della montagna? frase altrettanto importante: per noi la montagna è vita. Questo disegno di legge vuole dare questo significato alle popolazioni di montagna. La montagna è una realtà complessa. Come dicevo prima, c'è il fenomeno dello spopolamento, dato da tanti fenomeni che a partire dall'invecchiamento della popolazione e dalla diminuzione del tasso di natalità. Ma uno dei temi principali è la riduzione dei servizi; i giovani se ne vanno e di fatto si arriva alla

Facciamo un esempio molto semplice: se uno scuolabus deve andare a prendere i bambini nei paesi sottostanti delle valli, nel giro di 30 chilometri raggruppa tutti i bimbi; se invece deve andare a prendere i bimbi di montagna, quando ha finito di salire e scendere, i chilometri diventano 180. Questo significa tempo e denaro. Devo dire che il provvedimento era già fatto molto bene. Siamo intervenuti con alcuni emendamenti importanti. Ringrazio il senatore Paganella per l'intervento

sopravvissute nel tempo proprio perché vivevano in montagna, ma stanno subendo chiaramente quello che è il fenomeno dello spopolamento e, di conseguenza, il rischio

permessa allora di introdurre degli emendamenti per salvaguardare queste minoranze linguistiche. Ringrazio il Ministero per averli accolti. Tali misure riguardano la sanità,

anche per le minoranze linguistiche. È stato aggiunto inoltre un emendamento che dà maggiore contribuzione, sempre sul credito d'imposta, alle imprese che vengono istituite da giovani *under*

di solidarietà reciproca e per il mantenimento dell'economia produttiva e sociale necessita di una realtà cooperativistica. Volevo concludere

cuore e anima per dare le risposte che la montagna da tanto tempo attendeva e che finalmente con questo provvedimento vedranno la luce. *(Applausi)*.

quadrati su cui insistono i Comuni montani e parzialmente montani, che dunque rappresentano circa metà del territorio nazionale: basterebbe anche solo questo dato quantitativo considerare come una normativa specifica dedicata a queste realtà territoriali sia non solo necessaria, ma anche essenziale per la natura del nostro Paese. Da una parte, quindi, l'essenzialità e l'urgenza dovute alla sperequazione evidente che si registra da sempre e che è al centro del dibattito pubblico da anni, ma che dopo la legge n. 97 del 1994 non ha più trovato una efficace risposta nelle norme e nelle risorse via via stanziate, dall'altra la necessità di un quadro normativo che, al fianco della dimensione quantitativa del fenomeno, tenga conto anche degli elementi di merito che riguardano la grande questione delle aree interne e montane. Da questo punto di vista - e solo da questo - l'idea del Governo di proporre al Parlamento un testo di legge come quello oggetto dell'odierna discussione può essere raccolta come il segno di un'attenzione della quale dobbiamo farci tutti carico; purtroppo, il testo si caratterizza per carenze e lacune; è perlopiù fermo a dichiarazioni di principio che lo rendono non adeguato alla grande sfida che, nelle intenzioni, si incarica di affrontare. innanzitutto da un punto di vista giuridico, nella classificazione della fattispecie di Comune montano, questione alla base di ogni altra previsione normativa contenuta nel provvedimento in discussione: basta leggere l'articolo 2, "Classificazione dei Comuni montani", per comprendere come le previsioni normative contenute introducono elementi di complessità piuttosto che di chiarezza, che nella concreta applicazione della legge determinerebbero non pochi problemi. Di fatto, questo articolo rimanda all'adozione dei decreti ministeriali ogni indicazione sulla definizione e classificazione dei Comuni destinatari delle misure in discussione e lo fa indicando la strada di una sostanziale integrazione tra criteri di altitudine, pendenza e condizione socioeconomica. Un'integrazione tra criteri molto difficile e articolata, che rischia, nei suoi esiti finali, di restituirci una platea di Comuni disomogenea e distante, nell'applicazione della legge, dagli obiettivi originari; in altre parole, laddove i criteri geomorfologici fossero superati da una valutazione esorbitante della valutazione socioeconomica delle comunità locali, rischieremmo di avere una platea dei beneficiari delle misure di vantaggio previste del tutto impropria e inadeguata. di legge in discussione su questo rischio e su come porvi rimedio non si sofferma in modo efficace, come riportato anche in alcune delle audizioni svolte nel corso dell'*iter* parlamentare. Oltre a queste potenziali distorsioni, quello che si rileva da più parti è l'insufficiente investimento economico a corollario della norma già rilevato in Commissione dai colleghi Giorgis e Parrini tra gli altri. Non basta certo fissare obiettivi e auspici di sviluppo per rilanciare le aree interne, ciò che serve è certamente un grande investimento di risorse pubbliche. L'Unione delle comunità montane, nei suoi interventi pubblici di commento alla manovra in discussione e sul disegno di legge oggi in Aula, ha più volte parlato della necessità di risorse pari a un miliardo di euro, con un aumento del Fondo della montagna che oggi è fermo a 200 milioni di euro, un approccio che richiama il Governo a un'autentica presa di posizione che chiarisca le vere intenzioni: si tratta di una legge propagandistica, piena di propositi, oppure di un investimento reale e convinto per i territori montani? Ma alle osservazioni di merito normative ed economico-finanziarie che ho appena enunciato non può che essere affiancata una chiara e forte critica di tipo generale sul complesso delle politiche che il Governo ha messo in campo in questi anni e che impattano sulle aree montane. Siamo di fronte, infatti, a un testo che pone tra gli obiettivi di maggiore interesse quello di una tutela dei servizi pubblici come rilancio economico, lotta allo spopolamento e diritti alle persone. Lo fa ponendo in grande risalto il sostegno del diritto alla sanità e all'istruzione, il sostegno agli enti locali, cioè tutti quei settori e quei comparti che da due anni il Governo mortifica, con tagli e contrazioni di spesa e che, anche nel disegno di legge di bilancio in discussione alla Camera dei deputati, coerentemente continua a dimidiare. Sulla sanità pubblica e universalistica, come ormai noto, siamo al punto più basso del rapporto tra PIL e investimenti negli ultimi decenni e siamo in coda nei Paesi OCSE. Quando la Fondazione Gimbe ci dice che 4,5 di italiani rinunciano alla cura, quanti di questi 4,5 milioni sono anche cittadini e cittadine dei nostri territori marginali, delle aree interne e delle comunità montane? Il Governo, di fatto, svuota dotazioni finanziarie e servizi pubblici in questo comparto, danneggiando anzitutto i territori più marginali e orograficamente complessi. Mentre fa questo, con la mano destra pensa di poter annunciare al Paese, attraverso questa legge, una sanità di montagna, che suona come una promessa vana di fronte al fallimento del progetto di sanità territoriale, per il quale il Governo non si è mai speso, né ha saputo spendere i fondi del PNRR. Peraltro, lo fa prevedendo incentivi ai medici che accetteranno destinazioni montane, generando sperequazioni con quanti già oggi sono in servizio in queste aree del Paese, che non sarebbero assorbiti nelle novelle normative del disegno di legge in discussione, come già osservato in Commissione. Stessa distonia normativa e di risorse si registra sulla scuola, sia nella generale mancanza di investimenti sul comparto da parte del Governo, che con la manovra taglierà 5.600 docenti, sia, in particolare, in particolare, sul tema della scuola di montagna, che voi indicate nell'articolo 7. Va ricordato, infatti, come, anche in questo caso, il Governo negli anni sia già intervenuto con una riforma del dimensionamento scolastico gravemente penalizzante per i territori montani. I colleghi di maggioranza, in particolare quelli provenienti, come me, dalle aree interne, dovrebbero ricordare i nostri appelli a fermarsi allorquando, con l'approvazione della legge di bilancio dello scorso anno, furono introdotte nell'ordinamento le norme che hanno portato il numero minimo di studenti per il mantenimento degli istituti comprensivi e dunque dell'autonomia scolastica da 600 a 900 alunni. Un colpo alle comunità di montagna che, con l'applicazione della riforma, ha già determinato chiusure e accorpamenti, ma che negli anni, a regime, continuerà a mietere scuole. Ed ogni volta che una scuola chiude si spegne una comunità, come ha ricordato magnificamente Riccardo Milani nel suo ultimo bellissimo film "Un mondo a parte". che non si misura con le vere esigenze della scuola e delle ragazze e dei ragazzi che vivono in montagna, ma preferisce una dichiarazione di intenti su questa legge, dopo aver tagliato pesantemente con la riforma del dimensionamento. Infine, ma non certo ultimo in termini di importanza, legge si occupa di interventi a favore degli enti locali. Ed è persino ovvio, tenuto conto che alcuna nuova strategia sulle aree interne può essere immaginata senza un apporto decisivo delle autonomie Tuttavia, anche su questo settore non possiamo non rilevare il paradosso di un Governo che annuncia misure di sostegno ai territori, colpendo i medesimi con la scure di tagli molto ingenti. Parliamo di circa otto miliardi di tagli nel quinquennio, nel combinato disposto tra manovra in discussione e altri provvedimenti già assunti, compreso la manovra dello scorso anno, che mineranno pesantemente il normale funzionamento di Comuni e Province, scaricando disagi e carenze proprio su quei settori della scuola di montagna, della sanità di territorio, di sviluppo economico ed infrastrutturale che a chiacchiere si annuncia di voler tutelare e sostenere. Tutto questo nel mentre il Governo Meloni promuove nel Paese una riforma dell'autonomia differenziata, che fa proprio delle aree più deboli le vittime designate di un nuovo assetto costituzionale e di un e di un penalizzante riparto di competenze e risorse tra centro e periferie. Una norma sfascia Italia, una secessione dei ricchi, come ha detto Viesti, che aggrava sperequazioni e logora la coesione del Paese a danno del Meridione e delle aree interne. Sono queste le principali motivazioni che ci rendono scettici nella discussione di questo disegno di legge: non solo scettici, ma anche amareggiati, perché avvertiamo tutta la delusione di un'occasione persa su un tema tanto rilevante. Una legge sulla montagna sulle aree interne serve e l'intenzione del Governo di doverne fare un tema di discussione è e resta auspicabile. Purtroppo, a tale obiettivo non concorre il livello di inadeguatezza normativa e, soprattutto, di risorse che gli viene dedicata. La destra al Governo ha fatto delle aree interne e marginali del nostro Paese una bandiera di propaganda, secondo un principio di pratica politica che le è connaturato: aumentare ed esasperare i problemi e i disagi, senza mai dare una vera risposta. Purtroppo, anche in questo caso, anche con questo provvedimento, ha riconfermato tale consuetudine. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, signor Ministro, la legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, oggi in discussione (più tardi voteremo gli emendamenti ed esprimeremo il voto finale), è stata presentata dal Governo e dalle forze della maggioranza come un intervento tanto atteso,

Purtroppo, all'esito dei lavori della Commissione e visto il testo giunto in Assemblea, non sento di associarmi a questo coro entusiastico, ma - piuttosto - di dover rappresentare una grande delusione

Sgombero il campo da qualsiasi equivoco e possibile accusa di voler fare un'opposizione fine a se stessa e strumentale ed entro nel merito del provvedimento, come sono abituata a fare. Parto dai criteri di definizione di zone montane. Vi siete ostinatamente voluti fermare agli unici due criteri apparentemente oggettivi - il parametro altimetrico e la pendenza - come se siano, di per sé, criteri sufficienti a esprimere le caratteristiche di una zona montana. Avete fatto un'invasione di campo, invadendo l'ambito di competenza delle Regioni, come peraltro vi aveva già detto la Corte costituzionale, che aveva sancito espressamente il principio secondo il quale il

continua a lavorare insieme al CLEP per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Siamo in attesa di leggere, prima o poi, questi criteri. O forse non li leggeremo? Forse arriverà il Commissario e ce li sciorinerà belli e pronti. questo lo vedremo perché il futuro lo scriviamo insieme, o quantomeno ci speriamo. Il provvedimento in esame rappresenta, ancora una volta, una forma pratica e un esempio concreto di come questo Governo, da un lato,

economiche diverse da quelle ordinarie, degli agricoltori e dei silvicoltori, sul lavoro agile e sull'acquisto e sulla ristrutturazione di immobili. Pertanto, si salutano queste disposizioni dicendo che il Governo ha finalmente preso in mano la

alle autonomie, ai Comuni, continuare a tagliare le risorse agli enti locali e decidere, accentrando la spesa in maniera autoritaria, a cosa destinarle. Ancora una volta, abbiamo un Governo che da un lato dice di voler portare avanti il disegno sull'autonomia differenziata, dall'altro non fa altro che istituire e rafforzare organismi, misure e anche obiettivi di spesa e di programmazione della spesa in senso centralista, ma del peggiore centralismo, quello che non tiene conto neanche della voce dei territori, come non se ne tiene conto in questo provvedimento. La misura economica dell'intervento è davvero esigua e questo è un fatto che voi stessi avete dovuto riconoscere dicendo che è un inizio, una prima dotazione, una prima misura economica che mettete a disposizione, rinviando a un successivo provvedimento gli interventi interventi più cospicui e più importanti. Però, vede, signor Ministro, se gli interventi sono nella misura in cui li prevedete in questo disegno di legge, allora non ci siamo, perché se il mio obiettivo è quello di promuovere le zone montane, di limitare i disagi delle zone montane, di consentire alle popolazioni che risiedono nelle zone montane di superare i disagi esistenti o addirittura di attrarre persone, convincendole a trasferirsi nelle zone montane, allora in queste zone montane ci devo investire, ci devo mettere i soldi, ci devo realizzare le infrastrutture *(Applausi)*. Devo costruire strade, servizi, devo garantire che il personale dei servizi sanitari ci vada a lavorare, ma non con l'obiettivo che gli riconoscerò per un limitato periodo di tempo il doppio del punteggio, o darò ai professori e ai docenti un *bonus* economico se prendono in affitto un immobile, o addirittura se decidono di comprarlo, perché questa è una misura miope. Non solo è miope, ma è anche limitata nel tempo e soprattutto non convince nessuno, perché se io sono un docente, magari di prima nomina, forse sopporterò per i primi quattro o cinque anni il disagio di andarmi a trasferire una zona montana, ma poi perché ci dovrei andare a vivere? Perché dovrei decidere di stabilire là la mia vita *(Applausi)*, di farci una famiglia? Solo perché ho avuto un contributo al 60 per cento per l'acquisto di un immobile? Questo significa non dare valore alle cose, significa non investire sul territorio, significa non promuovere la cultura, significa non prendere davvero in considerazione i problemi delle economie locali. Significa, ancora una volta, decidere senza ascoltare i territori, perché i territori avrebbero detto altro. Avrebbero detto che per investire sulle zone montane non è necessario dire che si fanno gli accordi di programma o i partenariati pubblico-privati con i quali il gestore della rete delle strade si occuperà di manutenere le infrastrutture della telefonia mobile. Non funziona così e fin qua c'eravamo arrivati tutti: facile, facciamo un accordo di programma o comunque si accollerà i costi per gestire la rete della telefonia mobile e di Internet e poi con questa rete, che comunque sarà sempre il privato a gestire e a garantire, avremo la possibilità di promuovere il lavoro agile. Ma promuovere il lavoro agile non significa favorire la montagna, non significa far sviluppare la montagna. Significa trovare al solito un *escamotage*, un trucco, aggirare il problema. Allora, se investire sulla montagna significa semplicemente dare modo di sviluppare il lavoro agile, di fare la telemedicina, di dare un contributo economico per un brevissimo periodo di tempo, addirittura di dare un *bonus* cosiddetto bebè (fino a 5 milioni di euro però, non di più, attenzione) per chi nasce in questi territori,

le sperequazioni territoriali. Diversamente da quello che ha detto una collega che mi ha preceduto, non esiste una montagna "montagna" che sta in alto e vive con le economie della sua zona e una montagna bassa che invece vive grazie alle economie dei territori sottostanti. Questo non è il concetto di montagna, questo è il concetto di sperequazione territoriale, perché esiste una montagna alta,

non ci sono stati analoghi investimenti, dove per rifare la funivia che era crollata sono passati quasi dieci anni (forse è stata aperta ed inaugurata, ma fino a qualche tempo fa ma fino a qualche tempo fa era ancora ferma in attesa dei collaudi), e dove, a causa di mancanza di strade e di infrastrutture, grossi gruppi alberghieri e grossi investimenti economici non sono stati fatti. Dunque, o teniamo conto delle sperequazioni territoriali, del divario che esiste - esiste per scelte dello Stato negli anni che ci hanno preceduto - e agiamo per correggere e dare ai territori svantaggiati quello che serve loro, oppure tutte queste misure sono semplicemente dei palliativi che non risolveranno i problemi esistenti. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, tra poco più di un mese, l'11 dicembre, ricorre la Giornata mondiale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite ventun anni fa.

che entro pochi mesi questo provvedimento possa diventare operativo. Dico che questa è una speranza perché è abbastanza consuetudine in quest'Aula evocare e chiedere più risorse: tutti vorremmo risorse infinite e cerchiamo di dimenticarci

che potesse affrontare e dare la stessa dignità e gli stessi diritti di chi vive in città o in altri contesti alla gente di montagna. Sarò una inguaribile ottimista, ma credo che vada dato atto al Governo che pensare pensare di approvare una legge quadro sulla montagna significa non dividere la popolazione in cittadini di serie A e di serie B, ma riconoscere anche a chi vive in montagna il diritto ad avere un medesimo trattamento. Credo anche che le montagne siano un elemento essenziale perché occupano il 27 per cento della superficie terrestre, e certamente rappresentano un tratto fondamentale anche della nostra identità. La grande bellezza dell'Italia è anche la bellezza delle sue montagne; la montagna è quindi un tratto distintivo del nostro Paese, la culla di tradizioni secolari e di una civiltà speciale che ci ha contraddistinti. Tuttavia le montagne non stanno bene: ben prima che assumessimo consapevolezza delle gravi conseguenze del cambiamento climatico c'è stata una marginalizzazione della montagna, che ha causato anche uno spopolamento molto molto marcato. Recentemente, il presidente Mattarella ci ha ricordato, con un monito, che la montagna non può essere solo un immenso parco giochi e consumo dei flussi turistici, perché la regione di montagna è fatta di persone. È proprio a quelle persone che dobbiamo pensare, come alle tante che sono state travolte dagli eventi climatici avversi anche di queste ultime settimane. Avevamo e abbiamo il dovere di intervenire per tentare di spezzare quel circolo vizioso fatto di marginalizzazione, spopolamento, abbandono e ancora maggiore marginalizzazione. Come si prova a superare questa criticità? Innanzitutto attraverso una legge che rappresenta non la soluzione a tutti i problemi, ma sicuramente un buon inizio. Certo, poi serviranno i decreti attuativi. Tutti auspichiamo che ci siano maggiori risorse, ma con questo con questo provvedimento si segna un'inversione di tendenza e si compie un gesto concreto per fermare la marginalizzazione delle zone montane.

per dare una risposta a chi vive in montagna. Credo che vi siano alcuni interventi apprezzabili. Innanzitutto, le disposizioni contenute in questo disegno di legge si intersecano con tutta la produzione normativa che ha riguardato in questi anni le aree interne, con lo sviluppo e l'attenzione alla difesa e alla protezione del territorio e dell'ambiente, con la mole importante delle risorse del PNRR, impattanti anche sulle aree montane, con i futuri finanziamenti per i livelli essenziali delle prestazioni, che naturalmente devono riguardare anche gli abitanti delle terre alte.

Il disegno di legge, peraltro, prevede misure di incentivazione professionale per quegli insegnanti e quei medici che accetteranno di prestare servizio nei paesi di montagna; ricordiamo che attualmente non c'è nulla per le persone che si caricano questa responsabilità e svolgono un servizio nell'interesse del Paese. disegno di legge istituisce incentivi per le *startup* di giovani, per la residenzialità, per il lavoro a distanza. Mi piace citare, fra le misure contenute nel provvedimento, anche l'incentivo per la natalità, che è già stato evocato poc'anzi, che in qualche modo ha preceduto il *bonus* contenuto nel disegno di legge di bilancio appena presentato. Questo disegno di legge si occupa anche dei tribunali siti nelle zone montane, dei servizi di comunicazione, che spesso sono drammaticamente carenti, della valorizzazione dei pascoli e dei boschi, degli investimenti per ammodernare l'agricoltura e favorire la diversificazione, dei rifugi e dell'attività escursionistica. escursionistica. Vi è poi un elemento di metodo significativo. Ciascuno, man mano che va al Governo, si appassiona alle proprie proposte; poi i Governi passano e, quando non c'è una strategia d'insieme,

maggioranza e opposizione, dobbiamo sentirci addosso nei confronti delle future generazioni, come ci ha ricordato Draghi all'interno di quel piano sulla competitività che ha presentato in Europa. *(Applausi)*. Allora, il fatto che oggi il fatto che oggi al tema della montagna si affianchi una strategia per la montagna italiana dovrebbe essere visto da qualunque riformista, indipendentemente dalla tessera di partito che come un'assunzione di responsabilità. È un fatto positivo, al quale concorrere con ulteriori ricette e proposte, ma non limitandosi a chiedere più risorse, perché questo - ve lo ricordo - è un Paese profondamente indebitato e quei debiti li paghiamo noi e li pagano, in termini di competitività, di mancata crescita e di mancati posti di lavoro, le generazioni di oggi e di domani. *(Applausi).* Questo provvedimento non sarà perfetto, ma credo che in parte abbia ascoltato

che sia un passo avanti e che, anche dai banchi dell'opposizione, l'onestà intellettuale debba portare a riconoscere quando si fa qualcosa di buono. Per queste ragioni, annuncio fin d'ora il voto favorevole della sottoscritta e della collega Versace.

Se i soldi si investono dove servono, i risultati si vedono, tant'è che i risultati economici di questo Governo, che non investe neanche dove i soldi hanno dimostrato di portare frutti, si stanno vedendo. Abbiamo un PIL allo zero virgola, con prospettive per il futuro drammatiche con un'*austerity* che ci porta a un debito insostenibile, il quale invece era decisamente più sostenibile con misure di promozione della crescita e dello sviluppo del nostro Paese che sono sparite dai *radar*. Tornando però al merito di questo come dicevo, qualcosa di positivo si intravede. Ci sembra più una bellissima lettera di intenti che qualcosa di concreto su cui i nostri Comuni montani possano fare affidamento per il futuro, però almeno qualche spunto di riflessione, anche ascoltando gli altri, sembra che ci sia, come ad esempio la norma sul lavoro agile. Peccato che si fermi agli *under* 41: non si capisce per quale motivo ci debba essere un limite di età; si vede che gli anziani non vi piacciono o comunque non vi piacciono i lavoratori maturi, quelli sopra i cinquanta, che hanno pure difficoltà a trovare lavoro

lo capisco, ma provocatoriamente vi dico che non lo capisco, vogliate avvantaggiare solo chi trasferisce la residenza e non e non anche chi ce l'ha già, se la vuole tenere e non vuole migrare per andare a cercare il lavoro in una zona di pianura; anche questo è un mistero della fede. Non capisco perché limitare ai Comuni sotto i 5.000 abitanti (o, meglio, anche qui lo capisco). Anche tra i Comuni montani, per fortuna, ce n'è qualcuno sopra questo limite di popolazione; perché li penalizziamo, visto che notoriamente offrono qualche servizio in più e comunque aiutano a non spopolare le montagne? Ma va bene, magari poi nelle repliche avremo delucidazioni su questi limiti. Azzardo un'ipotesi: la coperta è corta e quindi bisogna ridurre la platea dei potenziali beneficiari. La coperta è sempre corta, quando

allentare un po' questa maglia troppo stretta secondo tanti, inclusa l'UNCEM, che è un interlocutore che ascoltiamo tutti molto volentieri, date le competenze competenze nel campo. Anche in questo caso, perché volete restringere la platea dei Comuni beneficiari? Perché la coperta è corta e quindi, se riducete il numero, magari riuscite a far bastare i quattro spiccioli che state mettendo in questo provvedimento. Vorrei ricordare a tutti noi in quest'Aula, e anche a qualcuno che magari ci ascolta da fuori, che stiamo parlando di

3.500 sono interamente montani e 500 lo sono parzialmente (ma

Parliamo spesso, per esempio, di una delle difficoltà: se qualche volta ci si prende l'ardire di avventurarsi su per le nostre montagne e andare a parlare con qualche abitante o amministratore, quello che lamentano più frequentemente è lo spopolamento dei servizi, in particolare sanitari. La nostra sanità è infatti un tallone d'Achille purtroppo da qualche tempo e ovviamente più ci allontaniamo dai centri cittadini, più tale fenomeno si manifesta in tutta la sua cruda realtà.

nelle valli del Piemonte, della Lombardia, ma anche nelle zone interne, collinari o montuose, dell'Umbria, arrivare a 50.000 abitanti significa raccogliere tre quarti della Regione, in alcune zone. E allora nelle aree densamente popolate dobbiamo fare affidamento, ovviamente, sul criterio della popolazione, ma forse, quando ci spostiamo nelle aree interne e marginali, dovremmo cominciare a ragionare nell'ottica dei chilometri quadrati da servire con determinati servizi che riteniamo essenziali, finché vogliamo continuare a considerarli

ragionano sul fatto di istituire classi scolastiche in deroga ai criteri attuali, oltretutto sulla base di organici già esistenti, quindi senza costi

Una banca - oltretutto sentita dai cittadini piemontesi del territorio, anche se adesso non è più prettamente "piemontese" - ha deciso ha deciso di chiudere lo sportello che aveva attivo storicamente in un Comune di poche centinaia di abitanti in una zona di montagna e persino di rimuovere l'apparato bancomat per erogare i contanti. Le Poste chiudono gli uffici nei piccoli Comuni; prima hanno diradato i servizi a due giorni o tre a settimana, adesso hanno annunciato, come penso sappiamo tutti, un piano di chiusura di quelli che ritengono servizi

infatti qualche vago accenno di spostamento dei conti da chi se ne va a chi rimane è stato fatto, le banche ci hanno sentito benissimo e hanno capito che forse non conveniva così tanto chiudere quello sportello. Quindi invito tutti, anche nell'ottica della maggioranza, che sta cedendo una quota azionaria di Poste Italiane, che fino a prova contraria è ancora una partecipata di Stato, a ricordare - non dico tirando l'orecchio, ma quantomeno suonando un campanello di avviso - a determinate imprese così importanti per la vita del Paese che hanno e devono avere un ruolo di responsabilità nei confronti dei cittadini italiani, soprattutto quando vivono nelle aree svantaggiate e quindi, se gli sportelli li vogliono chiudere, che li chiudano in una grande città,

con questo passaggio importantissimo, il disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane, legge quadro che - lo ricordo a quest'Assemblea - è stata fortemente voluta dalla Lega e portata avanti con la consueta competenza e soprattutto tenacia dal ministro Roberto Calderoli, passo avanti fondamentale verso l'obiettivo. Ricordo che le aree montane costituiscono il 54 per cento del territorio italiano, dove vivono 10 milioni di persone, con una produzione che è quasi del 15 per cento del prodotto interno lordo. La Costituzione italiana, poi, le richiama in modo chiaro ed esplicito all'articolo 44, in riferimento alla montagna, prevedendo che la legge disponga provvedimenti a favore delle zone montane, sancendo anche qui che l'ordinamento deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna, che rappresenta in Italia come in molte parti d'Europa - io direi anche del mondo - una diversità biologica e culturale straordinaria. Lo sviluppo dei territori montani costituisce un obiettivo di interesse nazionale, alla luce della rilevanza strategica delle zone montane, la cui crescita economica e sociale assume rilievo fondamentale ai fini della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, degli ecosistemi, delle risorse naturali, del paesaggio e soprattutto della salute. L'impegno del Governo e del Ministro è stato quello di mettere in campo una vera e propria strategia per la montagna, con risorse straordinarie, che valorizza e salvaguarda tutti questi concetti. È assolutamente necessario garantire sia maggior tutela dei servizi, a partire da istruzione e sanità, sia incentivi allo sviluppo e misure a sostegno del tessuto socioeconomico esistente, così da contrastare lo spopolamento e ridurre i divari territoriali. Fondamentale è anche una precisa definizione di cosa sia la montagna, per assicurare ai territori davvero montani tutto il supporto di cui c'è realmente bisogno. Questo provvedimento, finalmente, andrà a colmare una lacuna del nostro ordinamento. Con questa legge si punta a risolvere la problematica introducendo misure importanti a sostegno dei territori di chi abita e vive in montagna. Sappiamo che il territorio montano comprende attualmente circa 3.524 Comuni totalmente montani, poi ci sono 652 Comuni parzialmente montani, per un totale di 4.176 Comuni sui 7.900 del nostro Paese. In particolare, abbiamo due Regioni totalmente montane, la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, dove il 100 per cento dei Comuni è classificato montano. Partirei dal contenuto dell'articolo 11, un passo importante per la disciplina degli ecosistemi montani. In particolare, l'articolo in in questione reca disposizioni in materia di adozione di linee guida volte a individuare, recuperare, utilizzare in modo razionale e anche valorizzare i sistemi agrosilvopastorali montani, dalla promozione della certificazione delle foreste alla costituzione di zone associative tra proprietari e affittuari interessati. Il provvedimento prende anche in esame - e qui ringrazio la Commissione competente, fondamentale - la materia della tutela dei ghiacciai e dei bacini idrici fondamentali per la sopravvivenza della montagna e non solo, perché di lì scaturiscono i benefici idrici per tutto il Paese.

in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali. È prevista la possibilità di destinare una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane a interventi di carattere straordinario per la prevenzione e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e per far fronte alle criticità relative alla disponibilità

Richiamo anche l'articolo 13, che riconosce il contributo, sotto forma di credito d'imposta, agli imprenditori agricoli e forestali, ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie che esercitano la propria attività nei Comuni montani e che effettuano investimenti per servizi ecosistemici ambientali, benefici per l'ambiente e per il clima. Inoltre, viene consentito ai Comuni montani l'affidamento diretto dei lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile e di difesa dalle avversità atmosferiche, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, a coltivatori diretti, consorzi forestali, associazioni fondiarie che conducono aziende agricole ed ai gestori di rifugi. Qui ringrazio per aver preso in esame l'emendamento a mia prima firma, ma condiviso dai colleghi della Commissione agricoltura, che prevede che i requisiti per l'accesso ai benefici al credito d'imposta siano quelli di avere la sede legale nel Comune montano e di svolgere prevalentemente la propria attività nei Comuni montani, lasciando la possibilità di integrare il proprio reddito anche con servizi e attività effettuati fuori dal predetto territorio.

All'articolo 10 siamo riusciti a inserire un emendamento, con il quale, tra le finalità delle linee guida per la salvaguardia dei pascoli montani, si inserisce anche lo sviluppo dell'attività agricola, ed è questo, a mio avviso, il tema più importante. il tema più importante. Qui mi riallaccio al territorio del Piemonte, la Regione da cui provengo, che per un terzo è montano. È importante la definizione puntuale dei rifugi di montagna come strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e all'escursionismo e organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Si ribadisce anche qui che lo Stato e le Regioni autonome avranno la possibilità di stabilire le caratteristiche funzionali dei rifugi. Le condizioni peculiari dei lavoratori frontalieri e delle professioni di montagna sono state prese in esame benissimo. Nel cuore del disegno di legge c'è finalmente la norma che riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane, ferme restando le professioni di guida alpina, accompagnatore di media montagna, guida vulcanologica e maestro di sci, nonché quella di gestore di rifugio. La strategia nazionale per la montagna può individuare ulteriori professioni di montagna.

Infine, voglio concludere ricordando il valore di tutte queste norme, finalizzate a definire in modo organico e sistematico le politiche pubbliche destinate ai territori montani. Ci voleva chiarezza e chiarezza viene fatta, raccogliendo finalmente in un unico testo le varie misure a favore delle montagne, sulla base di criteri omogenei per la classificazione dei Comuni montani. Gli obiettivi principali sono sostenere le attività produttive esistenti, attrarre investimenti, fronteggiare il problema dello spopolamento, consentire alla popolazione residente di fruire di tutti i servizi essenziali, dalla scuola alla sanità, alla connessione, fondamentale, e alla mobilità, nonché promuovere l'agricoltura e la gestione forestale come un unico grande tema, anche tutelando e valorizzando il patrimonio culturale montano.

non disperdere l'importante patrimonio dei territori montani e tutelare le popolazioni dalle disuguaglianze. Anche questo è un grande tema sociale. Il disegno di legge è frutto di un cammino lungo e impervio, come sono le nostre terre alte. Cognetti scriveva che la montagna non è solo nevi e dirupi, creste, torrenti, laghi e pascoli; la montagna è un modo di vivere la vita, un passo davanti all'altro, silenzio, tempo e misura. Un passo dopo l'altro, grazie al lavoro del ministro Calderoli, lo dico qui a piene mani, diamo oggi finalmente alla montagna una legge quadro organica e strutturata, auspicando di cuore un futuro migliore a tutti coloro che vivono ogni giorno nelle zone montane. *(Applausi)*. Signor Presidente, colleghi senatori, con questo provvedimento ci stiamo occupando di una realtà estremamente importante del nostro Paese. Infatti, dei quasi 8.000 Comuni italiani, ben 3.500 sono montani, abitati da 7 milioni di persone. Abbiamo quindi tutti il dovere di affrontare il tema montagna con una visione ampia, non ideologica e attenta ai bisogni delle comunità che la vivono.

sulla volontà unanime di porre le condizioni per un'inversione di tendenza rispetto alla preoccupante dinamica di spopolamento in atto, non sono stati raggiunti.

si ridimensionano i servizi pubblici, a partire da scuola e sanità, e non si investono risorse sufficienti. Eppure, nel corso degli anni, anche alla luce delle drammatiche conseguenze di tanti eventi atmosferici, abbiamo visto cosa vuol dire disinvestire nella montagna e a cosa conducono la scarsa manutenzione idraulica, la poca cura degli alvei dei fiumi e la noncuranza per la forestazione. Per questo, bisognerebbe avere l'onestà di riconoscere, colleghi della maggioranza, che gli obiettivi contenuti nel disegno di legge avrebbero richiesto un'altra e ben diversa dotazione finanziaria, maggiore rispetto a quella prevista dal Fondo per lo sviluppo delle montagne Signor Ministro, lo dico a lei: ancora una volta, ci risiamo; si fanno delle leggi, ma ci si dimentica di metterci le risorse finanziarie adeguate. *(Applausi)*. Ancora una volta a prevalere è l'incoerenza l'incoerenza tipica tra i titoli e le parole del provvedimento e i fatti concreti, che semplicemente non ci sono. Rispetto alla classificazione dei Comuni montani siete stati sordi, non avete accolto i pareri resi durante le audizioni e le proposte emendative e siete rimasti arroccati solo su parametri altimetrici e di pendenza, senza affiancargliene altri di livello geomorfologico e socioeconomico, che sarebbe stato di fondamentale importanza considerare. Su un tema essenziale come la sanità non avete voluto procedere alla rideterminazione del fabbisogno di medici e specialisti nelle Regioni sul cui territorio insistono i Comuni montani, così come non è stata approvata la proposta emendativa, che pure avevamo fatto, che prevedeva un'iniziativa di promozione delle aggregazioni tra medici e pediatri nelle aree montane. Stessa cosa per la previsione di specifici investimenti per la telemedicina, in modo da favorire l'assistenza sanitaria e la medicina territoriale anche nelle zone che oggi sono fortemente penalizzate. Ancora, discorso analogo vale per le scuole di montagna, a proposito delle quali la maggioranza continua irresponsabilmente a ignorare i danni causati sul piano del diritto allo studio da un'impostazione meramente aritmetica, codificata dalle norme sul dimensionamento. Abbiate almeno la bontà, visto che non vi interessa salvaguardare i servizi pubblici essenziali, di risparmiarci misure *spot*, come gli incentivi alla natalità, che in un contesto del genere, mortificato come questo, rischiano di rimanere soltanto titoli da *brochure* elettorali. Dopodiché, poste di bilancio ben più considerevoli le avrebbero meritate la banda ultralarga, i servizi di comunicazione e trasporto pubblico, così come il turismo, su cui andrebbe fatta una seria riflessione, puntando sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale rispetto a certe dinamiche che rischiano di devastare la montagna, rendendola più un lunapark che una risorsa da preservare e valorizzare, come sarebbe giusto, pensando forme di promozione turistica che possono differenziare i flussi oltre la stagionalità. Sarebbero servite azioni di supporto per le attività commerciali, per le edicole ormai desertificate per i distributori di carburante, ormai anch'essi rarefatti. Sono tutti indicatori preoccupanti, che non possono essere ignorati, e non si può pensare di continuare con operazioni di leggero *maquillage*, che però per chi vive la montagna, parliamoci chiaro, hanno il sapore della beffa. Così le cose non potranno migliorare e le dinamiche che si estenderanno sempre di più saranno, per esempio, quelle che affliggono la provincia di Belluno, il Cadore, un'area conosciuta da ciascuno di noi per le Dolomiti, ma che conosce un fenomeno di spopolamento dovuto non solo alla denatalità, ma anche e soprattutto alla forte emigrazione, specialmente giovanile, fenomeno questo che, se non verrà affrontato con un'azione comune comune ed efficace, potrebbe portare al declino inesorabile di quel territorio. I numeri sono impietosi. Ho rivisto le proiezioni elaborate dall'osservatorio economico e sociale di Treviso e di Belluno. Nel 2031 la Provincia di Belluno potrebbe ritrovarsi ad aver perso, rispetto al 2021, circa 7.500 abitanti, di cui 2.550 solo nel Cadore e nel trentennio compreso tra il 2001 e il 2031 si passerà da 43.800 a circa 60.300 ultrasessantacinquenni, con il conseguente aumento della pressione dei servizi sanitari e socioassistenziali, con tutto ciò che ne consegue in termini di tenuta dell'offerta in un territorio che per la sua orografia pone anche problemi di accesso ai servizi. Ecco allora che non c'è altra via che investire risorse ed è qui che è ancora più ferma la nostra critica - per garantire i servizi e per adottare politiche di sviluppo in grado di garantire opportunità ai lavoratori e ai giovani, laureati e non. In concreto, nel pieno rispetto dell'ambiente, serve un intervento finalizzato allo sviluppo, per esempio, di una filiera corta del legno, 100 per cento *made in Italy*, dalla materia prima al prodotto finito. O ancora, non dimentichiamocelo, serve una più attenta politica rispetto alle concessioni per lo sfruttamento delle sorgenti e la commercializzazione delle acque minerali. Oggi abbiamo un oggettivo vantaggio per le multinazionali e una scarsa ricaduta per i territori. modo, occorrerebbe una fiscalità di vantaggio e in tal senso - voglio ricordarlo ancora una volta - questo provvedimento è proprio un'occasione mancata. Una fiscalità di vantaggio sarebbe stata necessaria per ammortizzare le diseconomie del vivere in montagna e abbattere quelle dovute alla burocrazia. Noi come Gruppo PD rivendichiamo l'approvazione di un emendamento sul sostegno finanziario locale: Regioni e Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, potranno definire ulteriori sistemi di agevolazione, riduzione ed esenzione da tasse, tributi e imposte di loro competenza. Resta il fatto che questo disegno di legge, lo diciamo con grande rammarico, è davvero un'occasione mancata per la montagna. Noi abbiamo provato a migliorare il testo. I nostri emendamenti miravano proprio a potenziare i servizi sociali, a dare incentivi alle giovani coppie, a sostenere la creazione d'impresa, a potenziare le infrastrutture di collegamento fisico o digitale e a favorire il recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato, che sappiamo quanto sia importante per poter vivere in montagna. Il nostro impegno, nonostante questa vostra legge ricca di annunci, ma povera di sostegni concreti e di risorse finanziarie, continuerà per inverare il dettato costituzionale rispetto alla specificità riconosciuta in Costituzione dalla montagna. Lo faremo seguendo le parole del presidente Mattarella che, riferendosi alla montagna, ha affermato che laddove la vita è più dura si fanno strada i valori più autentici della persona. A queste persone e a questa comunità noi abbiamo il dovere di offrire strumenti di sostegno e risorse, con la consapevolezza che tutelare il bene pubblico della montagna significa tutelare l'interesse generale del Paese. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi senatori, quello di oggi qui in Aula è un passaggio che possiamo definire storico, perché dopo trent'anni la montagna torna al centro dell'agenda politica. Come infatti hanno ricordato anche i colleghi che sono intervenuti prima di me, l'ultima legge sulla montagna risale al 1994. Oggi c'è dunque un passaggio storico che si fa grazie al Governo Meloni e anche all'azione del ministro Calderoli, che ha seguito l'*iter* insieme ai relatori, quindi alla collega Pirovano Pirovano e al presidente della 1a Commissione Balboni, che ha sapientemente condotto i lavori che hanno portato oggi all'approdo in Aula di questo provvedimento. Si tratta di corale, che non ha tagliato fuori le opposizioni, ancora una volta, nel senso che sono state raccolti, valorizzati e assorbiti tutti i suggerimenti che sono arrivati e tutti i contributi migliorativi; non c'è stata un'eliminazione un'eliminazione di tipo ideologico. Anzi, tutti gli interventi che miglioravano il provvedimento sono stati accolti senza veti in modo trasversale. Ricordiamo infatti che, degli ottantasei emendamenti che sono stati approvati,

Vorrei sottolineare un aspetto che spesso ci troviamo ad affrontare: quando si parla di montagna, si parla spesso di un territorio limitato e residuale, per cui le terre alte e le aree interne pagano spesso una visione una visione miope e stereotipata. In realtà - anche qui è già stato detto, ma ci tengo a ripeterlo - il 49 per cento del territorio italiano è classificato come montano,

assolutamente fondamentale e imprescindibile, quando si parla di futuro e di sviluppo della nostra Nazione. Credo che

politica, senza avere quell'approccio salvifico o eroico che c'è stato spesso in passato, come se le terre di montagna e le comunità che vivono in montagna dovessero essere soccorse soccorse o salvate. Dovremmo superare alcune storture ideologiche, perché la montagna si salva da sola. Le comunità che vivono in montagna sono in grado di cavarsela da sole, non hanno bisogno di paracadute o di

quel *gap* di opportunità che si è creato rispetto ad altre aree. Chiedono di poter liberare le proprie potenzialità e di farlo attraverso un percorso di valorizzazione condivisa. Questa non è ma si tratta di coesione; significa ridistribuire le risorse, anche tenendo conto che la montagna da sempre ha messo a disposizione tutta una serie di risorse che in realtà non le sono state restituite in maniera equa. Pensiamo alle concessioni idroelettriche e a quanta dell'energia prodotta rimane nei territori di appartenenza. di appartenenza. Un altro grande merito di questo provvedimento, oltre a mettere la montagna al centro dell'agenda politica, è quello di mettere l'uomo al centro della montagna. Credo che questo sia fondamentale rispetto a tutte quelle comunità che vivono la montagna ogni giorno. Una risposta chiara e forte deve arrivare soprattutto a chi vuole mettere la montagna sotto una campana di vetro, a chi vorrebbe, invece, che le aree montane rimanessero qualcosa di chiuso e intoccabile. Noi dobbiamo rispondere a tutte queste persone: giù le mani dalla montagna. In realtà, infatti, non c'è montagna senza uomo, senza le aziende, senza l'occupazione, senza i trasporti, senza le scuole, senza l'allevamento, senza l'agricoltura, senza le infrastrutture; in altre parole, non c'è montagna senza opportunità,

di un territorio a dettare le politiche, ma queste sono determinate, in realtà, dallo sviluppo di un territorio. Finalmente consideriamo strategico l'approccio al tema della montagna e infatti parliamo di «strategia nazionale per la montagna».

a 15 milioni di euro i fondi prima dell'istituzione del Fosmit, il fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, con la legge di bilancio del 2022.

sui punteggi nei percorsi di accesso ai ruoli dirigenziali per i medici e per il personale sanitario che accetteranno di lavorare in montagna; si aggiungono i crediti di imposta, sempre a loro riservati, a sostegno dei canoni di locazione. In tema di scuola, vi sono incentivi in termini di percorso delle carriere e crediti di imposta per i canoni di locazione. In termini di riordino fondiario, si prova finalmente ad affrontare e a risolvere la parcellizzazione che impedisce la nascita e il radicamento di aziende agricole solide e di dimensioni adeguate. Un ottimo intervento è anche quello per il contrasto dello spopolamento, con incentivi e misure economiche, come i finanziamenti e le agevolazioni fiscali, per chi decide di risiedere e lavorare nelle zone montane. C'è poi il contrasto del dissesto idrogeologico, anche attraverso la valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani.

corretta e armoniosa con la natura. C'è piena soddisfazione per il provvedimento in esame, che è un altro grande tassello nel percorso di riforma dell'Italia e un'altra grande vittoria del Governo Meloni.

si riconosce completamente nella sua esaustiva relazione. Quindi chiedo al Presidente, per la parte generale, di poter depositare il testo scritto della mia replica, Vorrei però mettere i puntini sulle "i" rispetto ad alcuni interventi, perché non ho mai apprezzato la politica del "fate quel che dico, ma non quel che faccio", che non funziona. non funziona. Alcuni dicono che non ci sono risorse o che ci sono poche risorse e che ce ne vorrebbero esattamente il doppio. Mi sta bene, io avrei voluto anche il quadruplo, se le avessi avute a disposizione; ma non le ho, quindi devo utilizzare quel che c'è. mia memoria solitamente è buona e quindi torno al passato: se le critiche rispetto alla mancanza di risorse mi vengono dai partiti che governavano nel 2021, quando a favore della montagna c'erano due o tre fondi per qualche milione di euro, mi chiedo perché non lo abbiano fatto nel 2021 questo intervento.

da dividere fra 2.000 soggetti che sono realmente montani, la fetta della torta avrà una certa dimensione, se invece il numero è più del doppio, verrà meno della metà della fetta che mi sarei aspettato. È inutile pensare, come si è fatto in passato, a tanti piccoli rivoli per accontentare tutti, perché alla fine non si accontenta nessuno e, soprattutto, manca un piano strategico e strutturale rispetto ai problemi dei Comuni della montagna. Lo dico perché anche in Commissione si è molto discusso rispetto ad altimetrie che non sono necessariamente classificabili come montane. Io abito a Città Alta, a Bergamo, a 362 metri, e ritengo

andranno affrontati e risolti con una legge *ad hoc* e non con interventi per la montagna. Non aiutiamo altrimenti né i Comuni montani, né tantomeno le aree marginali.

abbiamo calpestato l'autonomia di Comuni e Regioni e che proprio io avrei assunto questo ruolo. No, lei si sbaglia, io ho portato la legge, come parere in Conferenza unificata e Comuni, Province e Regioni si sono espressi tutti a favore della proposta di legge. La suddivisione del Fosmit richiede l'intesa fra tutte le Regioni.

La collega Pirro ha parlato di banche e poste. Condivido quello che lei ha espresso. Ho visto che è stato presentato un emendamento in questo senso e, come Governo, esprimeremo su di esso un parere favorevole, come mi auguro farà anche la relatrice. Credo, conclusione, che il meglio sia sempre nemico del bene; io mi accontento del bene di quest'oggi, che sono certo sarà sicuramente bene anche per la montagna e, quindi, per i miei amici della montagna.

9.0.150, 9.0.151, 10.157,

l'emendamento 1.150, che interviene sulle finalità della legge, è direttamente connesso all'impianto che questo tipo di provvedimento deve avere. Una semplice lettura del testo proposto dal Governo, varato poi dalla Commissione, e quello al nostro esame, fa comprendere la differenza dell'approccio rispetto alle finalità. Potremmo definire il testo che il Governo propone un testo sostanzialmente conservatore, di fotografia dell'esistente; invece noi vorremmo proporre un'impostazione più innovativa e riformista, capace soprattutto di tener conto del fatto che bisogna intervenire su due capisaldi che debbono essere fissati all'interno delle finalità e poi successivamente essere trasferiti all'interno del corpo giuridico. Questo evidentemente non avviene, ma ne discuteremo

della rete dei Comuni e delle autonomie locali nel nostro Paese, in particolare con riferimento ai temi delle aree montane. Il secondo aspetto è relativo al riconoscimento della peculiarità, delle prerogative e della specificità di questi territori in rapporto alla erogazione di quei servizi di prossimità e di quei diritti di cittadinanza che devono essere declinati sulla base delle caratteristiche di questi territori. Insomma, istruzione, trasporti pubblici, sanità e assistenza sono gli elementi indispensabili per assicurare qualsiasi tipo di futuro a territori di questa natura. natura. Dicevo che è indispensabile affrontare la questione delle autonomie, perché il testo di legge è, come è stato ricordato, un testo essenzialmente conservatore e centralista, che immagina un intervento dello Stato attraverso risorse che non ha più e attraverso competenze che sono state trasferite alle Regioni. È quindi inevitabile che, se vogliamo consentire ai territori di avere livelli di cittadinanza presidiati in maniera sufficiente, occorre intervenire rispetto ai temi che ho posto e rispetto alla seconda questione, che è quella dello sviluppo locale, attraverso il quale arrivano le condizioni di occupazione e di reddito che sono i secondi elementi fondamentali per i quali su questi territori si sceglie di rimanere o si può decidere di andare; questo inevitabilmente fa a pugni con la rete di poteri locali che oggi su queste realtà è disarticolata, differenziata e non ha la capacità di affrontare in maniera organica la complessità della modernità. Governo abbia deciso di non volere scientemente affrontare questo aspetto è uno degli elementi che fanno di questo provvedimento un disegno di legge monco e lo vediamo se andiamo ad affrontare il tema della platea dei Comuni montani, al netto delle osservazioni che ha fatto prima il Ministro, che mi permetto di confutare. Il tema Il tema della classificazione delle aree montane esiste in base alla legge n. 991 del 1952, ripresa successivamente dalla legge n. cristallizzata poi dalla legge n. 142 del 1990 e trasferita, poi, sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, nella competenza residuale esclusiva delle Regioni. Non è vero, quindi, che si sta parlando dell'esigenza di introdurre una nuova classificazione, ma è vero esattamente l'opposto, ovvero che si sta creando un ulteriore elemento di confusione nel tema della classificazione. *(Applausi)*. Del resto, ce lo ha confermato il Ministro dicendo che la coperta è corta e quindi bisogna diminuire la possibilità dei Comuni di stare sotto questa coperta, ma il problema non sarà risolto, anzi sarà acuito. Il tema vero, però, è la riorganizzazione e la modernizzazione di questa rete. Abbiamo proposto l'introduzione della comunità dei Comuni montani come elemento nel quale ci sia l'obbligo per i Comuni di lavorare insieme, di programmare insieme le risorse, di esercitare una funzione che non sia in competizione fra di loro, non in una dimensione di esaltazione del campanilismo che rischia di frustrare gli elementi della soggettività, ma come invece elemento di modernizzazione. Tutto questo tema, che rimanda inevitabilmente alla questione della riforma degli enti locali, viene espunto e quindi stiamo parlando di una cosa che non sta più in piedi e, per non affrontare questo nodo, semplicemente si decide di parlare di altro

all'interno di questa norma si sta pensando di dare la fantasmagorica cifra di 50 euro ad ogni… *(Il microfono Io vorrei anche concludere, se però il Governo fosse al suo posto, ma comunque non fa niente, evidentemente non sono degno di essere ascoltato dal Ministro competente.

lasciamo concludere il senatore Borghi. Senatore Zaffini, per favore, lasciamo concludere il senatore Borghi. RENZI Signor Presidente, per questo motivo, quindi, l'esigenza di dover intervenire in sede emendativa per sostituire l'impianto delle finalità corrisponde ad una esigenza precipua di dare una norma organica e non una norma manifesto a un pezzo significativo del territorio del nostro Paese.

il senatore Borghi voleva riscrivere tutte le finalità dell'articolo 1. Io mi sono limitato a proporre un aggiustamento, perché credo profondamente in quello che ha detto il ministro Calderoli: Calderoli: meglio il bene del meglio, in questi casi. Questo bene, però, non è stato accolto dalla Commissione. Dunque propongo quello che in questo provvedimento in genere manca, cioè di fissare dei princìpi fondamentali, che in rispetto alla normativa della gestione del territorio montano. In particolare, propongo di dire che è necessario il presidio umano in montagna. È necessario per conservare la montagna.

ma anche per la natura stessa, di cui la montagna è un contenitore, è necessario che la montagna rimanga su; e perché ciò avvenga c'è bisogno di persone che vivano in montagna, che la monitorino, che la utilizzino, che la salvaguardino. Pensiamo ai pastori, che una volta regimavano i corsi d'acqua, facevano le canalette nei pascoli e con questo salvavano i versanti. Dico questo anche perché noi sappiamo che, nelle sentenze che riguardano le attività umane in montagna, tendenzialmente il magistrato mette sempre davanti la conservazione della natura

"*al comma 1, dopo le parole:* «articolo 44, secondo comma, della Costituzione», *aggiungere le seguenti* : «e in coerenza con gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'UE»".

**Il Senato non approva**.

Signor Presidente, purtroppo è bastato attendere le votazioni sui primi emendamenti per constatare quello che durante la discussione generale

Grazie, Presidente. Presidente, già il senatore Enrico Borghi ha fatto la cronistoria delle diverse norme che hanno stabilito la classificazione dei Comuni montani e il senatore Martella insisteva in in discussione generale sulla necessità di appoggiarsi ai dati, in particolare demografici, perché questi sono fondamentali per stabilire il futuro delle popolazioni che risiedono in montagna. Anche qui va detto che c'è stata una richiesta di UNCEM di riprendere una serie di parametri che sono stati esclusi nel testo definitivo licenziato dalla Commissione e quindi provo a riproporli, facendo riferimento soprattutto al calo demografico degli ultimi due decenni, alla distanza e difficoltà di accesso a servizi pubblici essenziali, tempi di collegamento stradali e ferroviari con i centri urbani: tutta una serie di parametri attraverso i quali definire i Comuni che sono in difficoltà, in quanto in montagna, e di cui è necessario tenere conto. Poi, al quarto periodo, propongo di propongo di inserire le Regioni come proponenti perché qui, checché se ne dica, anche se la Conferenza Stato-Regioni ha dato il suo assenso in generale a questa norma (anche perché meglio una norma che niente, riprendendo sempre le parole del ministro Calderoli), le Regioni sono di fatto escluse da qualsiasi processo decisionale preparatorio e quindi chiedo che vengano tenute in considerazione, sia nella fase preparatoria, sia nella fase decisionale, prima di arrivare alla decisione finale.

dello spopolamento e le difficoltà che esistono in montagna, bisogna attenersi alla realtà: la realtà è che diminuiscono le persone, ma allo stesso tempo le necessità rimangono e, quindi, quando si fa una valutazione, gli elementi di distanza e la mancanza di servizi vanno tenuti presenti. L'emendamento è una fotografia della situazione e si dice di no: questa è una cosa davvero incomprensibile, per cui chiederei di riconsiderarlo.

2.6 e 2.7, poiché tengo a precisare che il tema verrà affrontato nell'ambito della riforma delle Province che attualmente è all'esame del Senato.

«sulla base di criteri volti a garantire il più ampio supporto informativo circa i diversi tipi e caratteristiche delle montagne,».

il tema sarà affrontato all'interno della riforma del TUEL.

Presidente, abbiamo cercato in tutti i modi di far capire che i criteri per la definizione di quelli che saranno i Comuni montani, e soprattutto di quelli che non lo saranno più, devono essere più elastici. Non ci si sul criterio altimetrico, sottovalutando gli altri parametri. Nell'emendamento 2.1 facciamo riferimento ai criteri geomorfologici, che possono essere legati alla pendenza e a particolari difficoltà che non sono dissimili dei Paesi che si trovano in alta montagna. In altri emendamenti abbiamo anche parlato di come sia importante tenere conto del criterio socioeconomico. In questo provvedimento invece sembra che si stia adottando lo stesso metodo che c'è stato per l'autonomia differenziata, ossia creiamo una *bad company*. Ci sono Comuni che, anche se si trovano qualche metro sotto il livello altimetrico,

Signor Presidente, questo emendamento non ha nessun impatto di carattere economico. Non si può a questo proposito né richiamare l'articolo 81 né

per quello che al Governo risulta, una definizione puntuale e attendibile di Comune montano. Noi prendiamo Noi prendiamo questa come una considerazione che si riferisce all'attuale normativa presente nel nostro Paese: la disciplina sui Comuni montani e sulle comunità montane, ad avviso del Governo, non è un criterio che può fornire una qualche indicazione. Allora, se è così, vorrei che su questo specifico aspetto vi fosse una risposta di merito da parte della relatrice o del Governo o da qualche esponente di maggioranza. Sinceramente, dopo ciò che abbiamo ascoltato in sede di audizione, dopo i rilievi che ci sono pervenuti anche in forma scritta, trovo incomprensibile il motivo che induce la maggioranza a respingere un emendamento che vorrebbe superare il criterio puramente fisico del del carattere altimetrico. Sappiamo benissimo - così ci avete detto anche voi - che il problema dello spopolamento e della carenza dei servizi riguarda realtà che soffrono e che hanno delle specificità dal punto di vista del calo demografico, dell'accesso a servizi pubblici essenziali, dei collegamenti. Allora perché respingere un emendamento che si limita ad ampliare i criteri sulla base dei quali definire le zone

l'errore di fondo di questo articolo. Signor Presidente, verrebbe da invitare il Governo e la maggioranza a rileggersi gli atti parlamentari. Infatti, la discussione che noi stiamo facendo il Parlamento della Repubblica italiana l'ha già fatta, ma l'ha fatta all'inizio dell'esperienza repubblicana, sulla legge n. 991 del 1952, cui promotore era un signore che si chiamava Amintore Fanfani, che peraltro era nato in un piccolo Comune montano della Toscana e che forse, seguendo l'applicazione dei meccanismi da alchimista del ministro Calderoli, non sarebbe più originario di una zona montana. Il presidente Fanfani all'epoca ebbe l'accortezza di affiancare all'elemento della fisicità quello dello squilibrio socioeconomico e demografico, proprio perché c'era un oggettivo rischio di disparità in una classificazione esclusivamente connessa a parametri di natura fisica, che rischiavano di introdurre all'interno del perimetro Comuni Comuni che magari avevano una oggettiva condizione migliorativa e di escluderne altri, semplicemente per un dato di natura fisica. Questa duplicità - rimando agli appassionati del settore - è stata ben definita da un presidente del CAI, il professor Salsa, nella differenza tra altitudine e altimetria, perché l'una rimanda a un concetto di scienza sociale e l'altra rimanda a un concetto di scienza fisica e, quindi, sono due questioni che hanno un diverso approccio. Questa impostazione è stata seguita in tutto l'ordinamento repubblicano, al punto tale che nel 1971, quando il legislatore introduce le Comunità montane, dice che questa cosa, che fino a ieri era di competenza dello Stato, da oggi (1971) diventa di competenza delle Regioni. Stiamo parlando di un'epoca in cui non si parlava di autonomia differenziata. Infatti le Regioni disciplinano le Comunità montane introducendo la classificazione dei Comuni montani e parzialmente montani esattamente per per consentire questo tipo di equilibrio. Si arriva poi alla legge n. 142 del 1990, che cristallizza il catalogo dei Comuni classificati montani e demanda successivamente, dopo la riforma del Titolo V, alla competenza esclusiva delle Regioni la classificazione dei territori. Ora qui si viene a dire che, siccome le Regioni hanno detto di sì in Conferenza delle Regioni, va tutto bene. Ma possiamo immaginare la reazione di un artigiano, di un commerciante, di un istituto scolastico che dalla sera alla mattina vedono escluso il loro Comune dai benefici previsti dalla legge per i Comuni montani? E immaginiamo che restino zitti e silenti e non adiscano ai provvedimenti di tutela delle loro garanzie? È evidente che qui ci sta infilando in un ginepraio in cui questa norma non sostituisce le normative precedenti, ma vi si aggiunge. quindi, di produrre più burocrazia, più ricorsi, più tempi e più confusione. E, quando sottolineiamo questo aspetto, lo diciamo perché è esattamente la differenza tra una norma manifesto e una norma organica. Se volete fare una norma organica, togliete questa cosa. Se invece volete andare sui territori delle Alpi a dire che avete cacciato finalmente i territori degli Appennini del Sud, che impropriamente hanno ottenuto i soldi in tutti questi anni, fatevi un attimino un esame di coscienza.

non ho compreso se il parere contrario della relatrice era riferito all'applicazione dell'articolo 81 o se si tratta di una questione più politica, relativa al rinvio alla riforma del TUEL. Non ho capito. *(Commenti)*. È la seconda, perfetto. Mi risulta difficile immaginare l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione su una proposta di carattere prettamente ordinamentale. Faccio proprio fatica a capire come questo sia applicabile. *(Applausi)*. Una volta esisteva la finanza innovativa e il ministro Calderoli adesso ci ha portato l'ingegneria istituzionale. questa discussione a nostro giudizio dovrebbe necessariamente tener conto del fatto che non si può continuare a rinviare, al giorno del poi, al mese del forse e all'anno del mai, la questione della riforma delle autonomie locali, di cui questo tema è sostanziale. Nei giorni scorsi il nostro Presidente della Repubblica ha ricordato, fra le quattro caratteristiche della nostra Costituzione, che una di esse - per le altre tre rimando alla lettura dell'intervento del presidente Mattarella; peraltro

Siccome all'articolo 5 si stabilisce che lo Stato uniforma il proprio ordinamento alle esigenze delle autonomie locali, immaginare che si possa fare una legge che riguarda i territori prescindendo completamente dalla natura, dalla funzione, dall'adeguatezza delle autonomie locali, significa fare una norma che, in spirito, non è repubblicana, ma è una norma più conforme all'idea conservatrice, da Statuto albertino, che dà l'idea di uno Stato immanente sovraordinato che pretende di intervenire con le proprie misure anche laddove queste misure sono di competenza del del sistema del reticolo delle autonomie locali. Insomma, con una mano ci venite a predicare le magnifiche e progressive sorti dell'autonomia differenziata, con l'altra cancellate la lavagna e riscrivete tutto in nome del centralismo statalista.

che occorre modernizzare la rete dei Comuni, che da soli non ce la fanno più? Voi non state portando in questo provvedimento un tema che ci avrebbe visti combattere con voi, e cioè il tema dell'autonomia tributaria, finanziaria, organizzativa dei Comuni per fare in modo che possano vivere delle risorse fiscali che i territori producono. Di Di questo non si parla, ma si parla sempre di rimesse statali, mancette ed elemosine che dall'alto scorrono verso il basso. Ma, se noi non ci poniamo il tema di come modernizzare questa rete, tutte le mancette che scivolano dall'alto verso il basso saranno inefficaci, non produrranno risorse, non produrranno risposte. Bisognerebbe, quindi, introdurre un meccanismo con il quale, da un lato, si riordina finalmente una platea, perché oggi nei territori montani c'è di tutto: i Comuni singoli che non fanno parte di esperienze associative, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane, i consorzi di bacino imbrifero montano, montano, gli enti parco, gli accordi di programma; c'è una sovrapposizione di poteri, di reti, di funzioni a cui corrisponde una debolezza strutturale ed insita di poter gestire la complessità dei fenomeni che ci sono in corso. Insomma, noi al posto di tutta questa foresta che frammenta il potere sui territori, abbiamo bisogno di un ente unico che aggreghi i Comuni e attribuisca loro l'esercizio associato delle funzioni e le competenze in materia di sviluppo locale. Per farlo, però, non abbiamo bisogno dell'attuale meccanismo in cui ogni Regione fa quello che vuole, con il risultato che una Regione ha le comunità montane, un'altra ha le unioni, un'altra non ha nulla, un'altra si inventa le Province, un'altra fa le Province a elezione diretta, un'altra torna indietro. questa grandissima confusione sotto il cielo, abbiamo bisogno di una operazione organica sull'intero territorio nazionale. L'introduzione di una comunità dei Comuni montani, che in maniera obbligatoria aggreghi i Comuni e attribuisca alle Regioni il compito di riordinare il potere locale, è una delle questioni fondamentali per la modernizzazione del sistema. Diversamente, continuiamo a pestare l'acqua nel mortaio.

Non è una proposta della minoranza cattiva, occhiuta, che vuole comprimere lo spazio di manovra. No, noi partiamo dal fatto che il Governo ha previsto la strategia nazionale per la montagna.

il Dipartimento retto dal ministro Calderoli, venga istituito un tavolo tecnico scientifico permanente per lo sviluppo della montagna;

dobbiamo calcolare il costo della realizzazione delle sedie, della scrivania e delle sale in cui si svolgono le riunioni per avere ammessi alla platea della discussione i nostri emendamenti, ditecelo. Altrimenti, spiegateci il motivo per il quale non volete entrare nel merito e vi nascondete dietro l'applicazione dell'articolo 81.

L'applicazione e il richiamo all'articolo 81 non possono essere fatti senza criterio. Lo abbiamo già sperimentato in sede di discussione sull'autonomia differenziata: si richiama l'articolo 81 e noi non siamo più nelle condizioni di pronunciarci su quelle che sono le vere scelte politiche. Ha ragione il senatore Enrico Borghi quando dice che qui si sta superando il limite della decenza. Si può discutere nel merito e si può bocciare un emendamento: ci mancherebbe. Non si può, però, richiamare in maniera così irresponsabile, così gratuita, una norma regolamentare. Questo non è possibile. Così come non è possibile presentare disegni di legge caratterizzati da una eterogeneità tale che diventa impossibile fare gli approfondimenti articolo per articolo. Allo stesso modo, diventa veramente uno sfregio al Parlamento al Parlamento e ai nostri doveri, prima ancora che ai nostri diritti, se si presenta un disegno di legge, si contingentano i tempi e diventa impossibile - come stiamo sperimentando in Commissione oramai da tempo - fare gli approfondimenti di merito. Il richiamo all'articolo 81 si inserisce in un contesto di complessiva svalutazione delle prerogative e dei doveri del Parlamento. di prendere sul serio questa lamentela. Non è una questione di indirizzo politico, di condivisione o adesione a una scelta: è questione di poter discutere nel merito le proposte che legittimamente vengono avanzate.

Signor Presidente, credo che l'emendamento colga un tema di fondo rispetto alla questione istituzionale che abbiamo definito. definito. Buona parte delle materie che riguardano sia i diritti di cittadinanza nei territori montani, sia il tema dello sviluppo di queste aree è già oggi di competenza delle Regioni.

Se poi parliamo di artigianato, commercio, forestazione, agricoltura o impiego dei fondi di coesione dell'Unione europea, anche queste sono già oggi tutte materie di competenza delle Regioni. Il Governo fa il seguente mestiere: spinge a tutta velocità l'autonomia differenziata. Vuole, cioè, che non esista più neppure una cornice di competenza concorrente fra Stato e Regioni, ma dice che le competenze sono tutte delle Regioni, e dall'altro ci viene a dire che la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si deve non si deve assolutamente interessare di tali questioni. Da una parte, stiamo facendo una legge dello Stato, con la quale a parole diciamo che risolveremo tutti i problemi; poi, nell'articolazione fondamentale dello Stato, abbiamo visto il Governo che non vuole impicci, niente tavoli, niente confronti, niente discussioni con gli enti locali o con i sindacati; tutte fumisterie, dicono di voler decidere loro. Certo, poi per dividere 100 milioni si fa anche piuttosto in fretta. Dal Dal punto di vista del coinvolgimento del Parlamento, però, zero: la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che è lì apposta, non deve essere coinvolta. siccome oggi siamo nel film del centralismo, la competenza sugli affari regionali non esiste. Poi chiederemo magari anche il parere del Presidente di questa Commissione se gli piace così tanto essere trattato in siffatto modo dalla sua maggioranza, ma in ogni caso c'è un'incoerenza di fondo, che dimostra una volta di più che questa è solo una norma manifesto; anzi, è solo una grida manzoniana per un po' di propaganda spicciola.

nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi dislocati nei comuni montani di cui all'articolo 2,

la riprova ne è il fatto che anche la maggioranza aveva presentato un suo emendamento, che ora apprendo dalla voce della collega Ambrogio essere stato ritirato. il Governo ha ritenuto di non accogliere neppure i suggerimenti che arrivano dalle file della sua maggioranza. Di che cosa stiamo parlando? Vedete, il tema della sanità nei territori di montagna sta letteralmente esplodendo, perché noi abbiamo l'incrocio di due congiunzioni complesse: da una parte, il tendenziale e progressivo invecchiamento delle popolazioni, che in termini di indice demografico è maggiore. Vedo che non interessa, ma chiederei di poter essere messo nella condizione di parlare.

di rispetto, se non di decenza, in quest'Aula dovrebbe essere assicurato, signora Presidente. Stavo cercando di spiegare… *(Commenti)*. Niente, siamo sempre alle solite. Io mi fermo. Non posso parlare in queste condizioni.

Stavo provando a spiegare i motivi per i quali questa vicenda è molto delicata, complessa e richiede un intervento. tratta di territori in cui vi è una percentuale di invecchiamento di popolazione maggiore rispetto ad altri territori. Sono territori nei quali l'accessibilità ai servizi è minore rispetto ad altri territori. E ancora: sono territori nei quali la possibilità di coprire gli organici di personale medico e paramedico è inferiore rispetto ad altri territori, perché non vi è una oggettiva condizione di prospettiva o di facilità. È più facile, infatti, fare carriera per un medico in grandi città, dove ci sono i policlinici, gli ospedali con un certo tipo di strutturazione e una qualità della vita e di accessibilità migliore e diversa rispetto alle vallate o alle zone periferiche. A ciò si aggiunga il fatto che stiamo facendo i conti anche con un ulteriore fenomeno, e cioè i territori del Nord, che confinano con la Svizzera, hanno lo svantaggio della competitività della vicina Confederazione elvetica. Non so se lo sapete, ma nel caso provo a spiegare che in Italia, in Piemonte, in Lombardia, al massimo un infermiere arriva a 2.000, 2.200 euro di stipendio al mese se fa i turni di notte o i festivi; se attraversa il confine con la Svizzera, prende di colpo 5.000 franchi, cioè più del doppio. Tutto questo naturalmente sta comportando un depauperamento delle strutture ospedaliere e della rete dei servizi. Noi abbiamo provato Noi abbiamo provato a proporre una serie di misure nella piena consapevolezza che non c'è la pietra filosofale su temi così complessi. La proposta che abbiamo provato ad avanzare prevedeva, per esempio, il fatto che l'attività prestata per almeno tre anni dai medici nelle strutture sanitarie e sociosanitarie venisse riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario, quantomeno per introdurre un meccanismo di incentivazione e di attrattività di questo tipo di elementi. Si proponeva altresì di introdurre un credito d'imposta nei confronti di coloro che acquistano in uno dei Comuni montani un immobile ad uso abitativo, per poter venire in quei territori a svolgere quel tipo di funzioni. Un altro tema molto complicato la scomparsa progressiva dei medici di base su quei territori. Ci sono infatti Comuni in cui i medici di base semplicemente non ci sono fisicamente più. Ecco, rispetto a questo sforzo di entrare nel merito, omettendo tutti

a un emendamento della collega Maiorino, che noi naturalmente voteremo, che è la descrizione di una condizione piuttosto insipida. Ci si viene a dire che le Regioni e le Province autonome ad invarianza di costi, senza incidere, eccetera, possono prevedere particolari forme, ma questo lo possono già fare oggi. Stiamo facendo, cioè, una norma per dire alle Regioni che possono fare cose che già oggi potrebbero fare. E, se non lo fanno, evidentemente non hanno bisogno di una norma in cui diciamo a qualcuno che può fare una cosa che non sta facendo. Anche in questo caso, si dimostra che stiamo votando una legge vuota.

perché - come è noto - l'adeguata assistenza sanitaria è determinata dal fabbisogno dei medici specialisti che sono presenti. richiamo ulteriormente i dati contenuti nelle banche dati del Ministero della salute e delle Regioni che comprovano le problematiche di carenza dei medici di medicina generale nei territori montani e rurali. Questo è un tema di grandissima attualità e di grande bisogno, e non penso soltanto alle vallate alpine da cui provengo. Vedo il collega Licheri potrebbe tranquillamente parlare e spiegare cosa succede in Sardegna su questi temi. Parliamo di un territorio che probabilmente non verrà più classificato montano se questa legge diventerà operativa, ma i problemi resisteranno tutti, anzi si acuiranno ulteriormente. Stiamo provando ad intervenire in uno spirito di naturale discussione parlamentare, che su questi temi ci fossero una capacità, una volontà, uno spirito di dialogo da parte della maggioranza, che invece prosegue tetragona a dare i pareri contrari a tutte le proposte della minoranza, addirittura a bocciare, quando ci sono questioni salienti, le proposte dei propri parlamentari di maggioranza e, se proprio deve chiosare, fa qualche piccola concessione sostanzialmente ininfluente rispetto all'impianto complessivo. Con vorremmo proporre che i medici di medicina generale che esercitano la professione nei Comuni montani avessero il diritto a ricevere una premialità economica determinata in maniera proporzionale al numero dei residenti assistiti e alle difficoltà di accesso ai servizi sanitari nel Comune montano di riferimento. E chiediamo che la Regione, con apposito regolamento, istituisca un fondo dedicato alle risorse necessarie per l'erogazione della premialità. Si tratta di una questione complessa, e me ne rendo perfettamente conto, perché si tratta di incidere sulla retribuzione degli addetti sanitari. Delle due l'una, però: o continuiamo a mantenere l'attuale massificazione della retribuzione e, quindi, non consentiamo una condizione di attrattività di determinati territori; oppure, esattamente come accade in altre circostanze e per altre forme professionali, prevediamo un incentivo specifico per questi territori. Signora Presidente, lei sa che in questo momento, mentre noi stiamo discutendo, ci sono 45 nostri poliziotti che stanno curando il nulla in un centro in Albania e che giustamente vengono maggiormente retribuiti, perché hanno un'indennità di missione per quel tipo di attività. *(Applausi)*. Come è possibile che in questo Paese si possa giustamente dare un'indennità di missione a dei poliziotti che stanno controllando il nulla in Albania e non si possa discutere di un'indennità aggiuntiva

zone montane. Tutti noi - ma soprattutto chi abita in quelle zone - sappiamo che, tra le specificità, ci sono necessariamente parametri diversi per il numero degli abitanti e, conseguentemente, il numero dei bambini. Se questi parametri, oggi in vigore

un organico aggiuntivo che era stato dato dalla Buona Scuola nel 2014 per le necessità delle scuole. Usate quell'organico, anziché tagliarlo,

Per ogni bambino che trova spazio in un nido, ci sono almeno tre persone che rimangono a vivere in montagna, quasi sempre per tutto il periodo dell'anno scolastico fino a quindici anni.

creando asili nido e luoghi in cui le persone e i bambini possano rimanere, tenendo conto delle specificità. Non possiamo non dire che ci sono delle specificità rispetto alle aree metropolitane,

quindi cercato di fare un lavoro supplementare per capire se non sia opportuno valutare la fattibilità di misure diverse, proprio in base al tipo di Comune. Quindi, potrebbero essere dagli aiuti diversi per la conciliazione famiglia-lavoro. Questa è la motivazione dell'invito al ritiro. Cercheremo di valutare altre soluzioni, ovviamente non al Senato, ma nel prosieguo dell'*iter* del provvedimento o con altri provvedimenti, perché il tema è di fondamentale importanza. [BORGHI Presidente, vorrei ringraziare sia la collega Rando per avere portato all'attenzione dell'Assemblea questo tema, sia la relatrice nel suo sforzo di cercare di venire incontro alle istanze, ma che sostanzialmente conferma l'impossibilità di poter procedere in termini di risposta concreta. Credo che questo elemento faccia venire a galla una volta di più il difetto di fabbrica che cercavo di descrivere in precedenza: non non aver voluto affrontare il tema del dimensionamento, dell'aggregazione e della integrazione del lavoro comunale in quei territori inevitabilmente fa scontare una incapacità di fornire una risposta su un tema così complesso. Anche sulla base di un po' di anni di esperienza accumulata, potrei dire che per un sindaco aprire un asilo nido in un Comune montano significa affidarsi alla cabala, perché significa aprire una struttura che ha forti oneri gestionali, molto consistenti, che non ha nessuna garanzia dal punto di vista della prosecuzione dell'attività, perché la curva demografica è quella che è. Inoltre, il costo di questo tipo di impostazione grava esclusivamente sul bilancio del proprio ente, con il paradosso - che si realizza non solo per gli asili nido, ma per tutto il *welfare* - che i Comuni che hanno fatto scelte in termini di *welfare* e di erogazione di servizi vengono doppiamente penalizzati, perché è totalmente a loro carico il peso dell'erogazione del servizio del servizio e perché il Governo, nella fattispecie quest'anno, introducendo il meccanismo dei tagli lineari, va a colpire i Comuni che hanno la spesa storica sociale più alta, quindi sono due volte penalizzati.

Penso che si debba considerare con grande attenzione questo aspetto, senza rinviarlo *sine die*. Se non affrontiamo il modo in cui si organizzano, si pianificano, si finanziano e si sostengono gli asili nido in questi territori, noi semplicemente di asili nido non ne avremo e quindi cristallizzeremo una condizione di subalternità in termini di diritto. Vedete, colleghi, serve a poco dare la mancetta di 50 euro alle famiglie che hanno la possibilità di dare vita ad un nascituro, se poi non si consente loro di avere una serie di servizi fondamentali. E questo è uno degli indicatori fondamentali che le famiglie vanno a cercare, se decidono di rimanere o di venire, perché, se uno non ha un asilo nido, semplicemente in un Comune non ci sta più e se ne va dove quell'asilo nido c'è. Non affrontare questo tema, nonostante la buona volontà che ho sentito in quest'Aula da parte della relatrice, è ancor più e una volta di più la dimostrazione che è una legge vuota.

è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. *(La seduta**, sospesa

una nuova finestra") Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, comunico che la seduta è sospesa fino alle ore 18. *(La seduta, sospesa

La seduta di oggi, senza orario di chiusura, prevede il seguito della discussione del disegno di legge sulla valorizzazione delle zone montane. Le dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento avranno luogo domani mattina, a partire dalle ore 9,30. Seguirà l'esame degli argomenti già iscritti in calendario e alle ore 15 si terrà il *question time*, con la presenza dei Ministri dell'interno, del lavoro e dell'università. Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei decreti-legge sul contrasto alla violenza contro gli operatori sociosanitari e salva infrazioni. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su quest'ultimo provvedimento, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto sulla fiducia, alle quali seguirà la chiama. Restano confermati gli altri argomenti già previsti. Nella settimana dall'11 al 14 novembre il Senato terrà seduta nelle giornate di lunedì 11, a partire dalle ore 16,30, e martedì 12, a partire dalle ore 10, senza orario di chiusura. Il calendario della settimana dal 19 al 21 novembre è integrato con la discussione dalla sede redigente del disegno di legge sul potenziamento dei controlli sanitari per il Giubileo 2025. Nella settimana dal 26 al 28 novembre sarà discusso il decreto-legge in materia di misure economiche e fiscali.

Presidente, è stato inizialmente assegnato alla Camera in data 23 ottobre e poi il Governo lo ha richiamato. Chiedo

Le colleghe e i colleghi di opposizione hanno chiesto, come era corretto che fosse, un *iter* chiaro che consentisse ai tanti mondi esterni al Parlamento di partecipare al confronto necessario.

va dalla furbizia alla ricerca di scorciatoie da parte del Governo. Il Governo ha annunciato oggi che quel provvedimento, presentato al Senato dopo che era stato presentato alla Camera, resterà in

anche in maniera irrispettosa verso il Parlamento, un emendamento che riprende lo stesso decreto-legge. Troviamo che ciò sia un'umiliazione per il Senato, signora Presidente,

così come accade nella vita, la mancanza di lealtà tra noi è causa di fallimento, in questo caso delle istituzioni stesse. Quando le istituzioni

So che in questa fase siete concentrati sul provvedimento in materia di regolamento per gli animali, ma la fedeltà si dà

Presidente Rossomando, le chiedo davvero di richiedere al presidente La Russa, per conto del Gruppo Partito Democratico, di fare di tutto per far sì che che le audizioni si svolgano fino a quando il decreto-legge non sarà stato ritirato dal Governo, perché se il Governo ritira il decreto-legge, allora il dibattito si sposta alla Camera sull'emendamento, ma se il decreto-legge è in vigore noi pretendiamo, presidente Balboni, Balboni, una risposta su quelle audizioni. Questa mattina - e chiudo, presidente Rossomando - in Commissione politiche dell'Unione europea l'opposizione è intervenuta - lo dico perché si lega a questa vicenda accaduta in 1a Commissione Commissione - contro la proposta del senatore Borghi per un'indagine conoscitiva sui magistrati italiani per le questioni relative alla conformità con il diritto dell'Unione europea. Ora, se un magistrato italiano,

disapplica la normativa nazionale per contrasto con il diritto dell'Unione europea, non è eversivo, colleghe e colleghi della maggioranza *(Applausi)*, ma sta semplicemente adempiendo al suo dovere, riconoscendo il principio del primato del diritto europeo rispetto al diritto nazionale. Perché se non è così, signora Presidente, se è il Governo italiano che decide al posto del Parlamento di fronte a un dubbio interpretativo di diritto dell'Unione europea o di fronte a un giudice che chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, quindi se tutto questo voi non lo consentite, allora significa davvero che confondete il governare con il comandare, ma governare non significa comandare *(Applausi)*, significa rispettare le regole democratiche e le regole dello Stato di diritto. Su questo non vi consentiremo di rompere ancora, presidente Balboni, il patto di lealtà che consente a quest'Assemblea di essere quello che ancora per noi è: il luogo solenne della democrazia italiana.

che gli interventi sull'ordine dei lavori possono essere richiesti solo dal Capogruppo; altrimenti, se sono per fatto personale, vanno rimandati a fine seduta. Naturalmente, essendo stato chiamato in causa il Presidente di Commissione, è ovvio che può e deve intervenire. Quindi le chiederei

*(FdI)*. Signora Presidente, intanto desidero dire a lei e a tutta l'Assemblea che non intendo raccogliere gli insulti che ho appena ricevuto dal presidente Boccia,

E lei non si deve permettere di offendere un Presidente di Commissione che rispetta e applica il Regolamento, caro signor Boccia. *(Applausi)*. Impari lei il rispetto delle istituzioni. Sulle audizioni c'è stato un confronto sereno e pacato in Commissione; il Capogruppo del suo partito, il senatore Giorgis, mi ha riconosciuto la correttezza della procedura con cui ho operato. Sulla richiesta di audizioni la Commissione ha votato e, fino a prova contraria, in democrazia è la maggioranza che decide e non è la minoranza che impone alla maggioranza quello che vuole. Dopodiché, ho riconosciuto alla correttezza del capogruppo Giorgis che la questione era squisitamente politica e che su una questione politica era giusto che ci si esprimesse politicamente. Non discuto le ragioni dei Gruppi di opposizione; discuto sul fatto che alla fine la questione si era ridotta al punto se fare o non fare le audizioni. La maggioranza della Commissione ha ragionato in questi termini,

Quindi mi sono anche impegnato su un piano personale, come Presidente - perché, a differenza di lei, io il rispetto delle istituzioni ce l'ho quando arriverà il testo dalla Camera, troveremo il modo di farle, le audizioni, ma su un testo chiaro, preciso e votato dalla Camera e non sulla previsione o sulla presunzione di un testo che non sapremo quale sarà.

di richiamare il presidente Boccia al rispetto dei colleghi, persino dei suoi avversari. le interpretazioni sono assolutamente libere. Intanto lei ha esposto la sua ricostruzione dei fatti, che è a disposizione dell'Assemblea. Mi è parso che fosse stata fatta una

Signor Presidente, farò alcune considerazioni, anche alla luce dell'intervento del presidente Balboni, e qui mi rivolgo a lui ovviamente per il tramite della Presidenza. Proporre in modo magnanimo audizioni sul decreto-legge che dalla Camera verrà trasmesso al Senato, dopo l'introduzione di un emendamento che ancora non c'è

È evidente che le audizioni servono per predisporre testi emendativi. Una volta che il testo sarà stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, non potrà essere più modificato, perché sappiamo benissimo che i tempi per una terza lettura non ci saranno. Quindi quelle audizioni non avranno nessun significato rispetto all'*iter* del provvedimento. Primo elemento. Secondo elemento: il presidente Balboni ci ha informato (ma la cosa era già nota) che non esiste ancora l'emendamento del Governo che riprende il testo del decreto Paesi sicuri e lo inserisce in un altro provvedimento. È stata un'anticipazione del Governo, che ha manifestato la sua volontà. Fino a quando ciò non accadrà e il decreto alla Camera non sarà completato, l'*iter* del decreto del 28 ottobre deve continuare come nulla fosse, perché nulla c'è. Al di là del contenuto politico del decreto, c'è una questione di rispetto delle istituzioni e degli *iter* del Parlamento, che non capisco perché debbano essere stravolti. È già avvenuto molte volte, in molte legislature, che un decreto venisse recepito come emendamento in un altro testo. Ma l'*iter* è sempre stato molto lineare: fino a quando non c'era il provvedimento emendativo, l'altra parte analizzava il testo del decreto come se nulla fosse, perché nulla c'era. Termino riprendendo le parole del presidente Boccia. La frase del presidente Balboni «siamo la maggioranza e facciamo quello che vogliamo» rappresenta molto bene la differenza che c'è tra governare e comandare.

Aggiungo la parte relativa a quanto è di mia conoscenza, rispetto a quanto è stato detto prima dal presidente Boccia. Per quello che riguarda la trasfusione del decreto, nulla osta da parte del Gruppo Lega, perché si tratta di una cosa molto frequente. Non capisco lo sdegno; tante volte, tante volte, almeno per quanto riguarda le questioni economiche, quando il ministro era Gualtieri i decreti di materia economica iniziavano e poi si trovavano trasfusi o inseriti, in certi casi fino a tre decreti in uno. meraviglia e questo spregio del Parlamento. Viceversa, per quello che è stato detto stamattina in Commissione politiche dell'Unione europea, io scuso il presidente Boccia, perché probabilmente si informa su «la Repubblica» e quest'ultima probabilmente si informa da qualcuno che dice cose sbagliate; quindi evidentemente può essere che sia stato tratto in inganno. Ovviamente io non ho chiesto nessun tipo di indagine conoscitiva nei confronti dei magistrati, cosa assolutamente incredibile. Guardatevi i Resoconti, così poi dopo potete valutare se sia vero o meno. Io ho chiesto un'analisi conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che non è un'indagine sui magistrati, ma è un'indagine che dovrebbe preoccupare tutto questo Parlamento. Voi capite che, se noi facciamo un provvedimento di legge (che sia proveniente da un decreto o da un disegno di legge) e non si capisce se è un testo definitivo o è un testo che può essere disapplicato da un magistrato, a me non interessa cosa decide il magistrato singolo, mi interessa la procedura; mi interessa la possibilità che un magistrato possa disapplicare una legge emanata da questo Parlamento sulla base del contrasto non solo

che questa situazione, che mi sembra molto pericolosa, venisse analizzata e spiegata da dei giuristi. Magari ci dicono che è normale così; a questo punto ne siamo a conoscenza e ci sappiamo regolare. Magari ci dicono invece che altri Paesi, come mi sembra di tutta evidenza, stanno facendo quello che vogliono. La Germania manda la gente in Afghanistan, tanto per dirne una, e non mi sembra esattamente un Paese tranquillo e sicuro. Evidentemente forse l'Unione europea è differente in Germania rispetto all'Italia. Allora a quel punto che noi si sappia se si devono fare delle modifiche ed è colpa nostra perché siamo meno sovrani rispetto alla Germania oppure se invece le cose stanno così, e allora, a quel punto ci sappiamo regolare tutti. Quindi nessuna cosa contro i magistrati, in nessun caso. si chiede un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, che mi sembra più che necessaria. È stato quindi male informato, deciderà l'Ufficio di Presidenza della 4a Commissione se sia il caso di sentire o meno degli esperti. Dal mio punto di vista più informazioni ci sono e meglio è per tutti. se l'Ufficio di Presidenza deciderà che non è il caso di sentire degli esperti, che potrete indicare anche voi, me ne farò una ragione. Quindi nessuna eversione, nessun problema.

senza avere bisogno di un'indagine conoscitiva di altri esperti. *(Applausi)*. Il principio del primato del diritto dell'Unione europea sul diritto nazionale è un tema acquisito non solo dai giuristi, ma anche dai legislatori. Esiste

ha a che fare con una normativa nazionale, anche successiva, è tenuto a disapplicarla. Questa non è eversione, ma adempimento *(Applausi)* di ciò che significa essere nell'ordinamento costituzionale italiano ed europeo. Se un giudice nazionale davanti a un dubbio interpretativo fa un rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte del Lussemburgo, questa è una facoltà per il giudice nazionale, ma è un obbligo per il giudice di ultima istanza. non lo fa, scatta la procedura di infrazione, cioè la responsabilità dello Stato italiano. Possiamo fare tutte le indagini conoscitive che vorremo, ma non avrà un risultato diverso da quello che le sto dicendo, senatore Borghi, come lei sa benissimo. Ecco perché presentare un emendamento, con un atto avente forza di legge, non ha alcun valore giuridico. Allora il tema è politico e si riassume in questo, senatore Borghi: se una parte della maggioranza accetta o meno il principio del primato. del primato. Se non lo accetta, la risposta non è un'indagine conoscitiva sulla gerarchia delle fonti, ma il fatto che una parte della maggioranza si assumerà la responsabilità di dire che non vuole stare in Europa. *(Applausi)*. Abbiate il coraggio di dire le cose fino in fondo, non appellatevi a criteri giuridici quando la scelta è politica. Questo è quello che abbiamo detto oggi in Commissione e mi fa piacere averlo condiviso insieme a voi in Assemblea. Signora Presidente, vorrei riportare il tenore della nostra discussione sul fatto che è stato sollevato in precedenza e che dal punto di vista politico, merita di dover essere sottolineato. Noi abbiamo assistito intanto ad un elemento procedurale indiscutibile. In sede di Conferenza dei Capigruppo, il Governo si è presentato e ha annunciato formalmente che non intende dare corso alla conversione all'interno del Senato del decreto-legge ribattezzato Paesi sicuri e che intende trasformare il suo contenuto in un emendamento ad un provvedimento che oggi è allocato alla Camera. a me interessa cogliere il punto politico di questa vicenda. Capisco che nell'enfasi della comunicazione abbiamo tutti la memoria del pesce rosso,

Il Ministro dell'interno si è presentato poche ore dopo il Consiglio dei ministri nella cosiddetta terza Camera della Repubblica, cioè il salotto di Bruno Vespa, ad illustrarci con un'enfasi da questurino che finalmente avevano trovato la soluzione per la quale c'era giuridicamente la possibilità di classificare 19 Paesi come Paesi sicuri. E quindi da questo momento sarebbero riprese le attività di trasbordo, trasporto o definitele come volete, di migranti in Albania, perché era questo l'elemento giuridico che vi stava in quel momento a cuore, cioè tentare disperatamente di tornare indietro da una brutta figura planetaria che avete fatto. Ora, che cosa sta accadendo? Noi ci saremmo attesi, visto che avevate tutta questa enfasi, questa *vis* polemica, questa ansia di regolare i conti con chi, a vostro parere, a vostro giudizio, a vostra definizione, vi aveva impedito di mettere in atto una procedura per mettere in sicurezza i nostri confini, che voi per primi vi alzaste in quest'Aula e rivendicaste il vostro diritto-dovere di sostenere qui quello che Piantedosi, Nordio e la Presidente del Consiglio hanno detto *coram populo* e invece no.

una situazione che domani cercheremo di chiarire con il ministro Piantedosi - che ogni tanto, oltre ad andare da Bruno Vespa, si deve degnare di venire qui a spiegare come mai in Albania ancora non c'è nulla e come mai continuiamo a buttare soldi nella fornace e come mai tutto questo non sta funzionando - ora voi state tornando indietro. Il motivo, al di là degli elementi di natura procedurale, è che avete in primo luogo paura del rinvio oggi annunciato alla Corte di giustizia europea, perché sapete benissimo che un pronunciamento di quella Alta corte smentirebbe definitivamente tutta questa narrazione. La conferma arriva dall'intervento del collega che ha il mio stesso cognome, ma che la pensa esattamente all'opposto rispetto a me, il quale ha confermato che avete paura del pronunciamento della Corte di giustizia europea e sapete benissimo che questa bloccherebbe definitivamente ogni valore giuridico di quel decreto che ogni giorno che passa perde qualificazione. Cosa dovete fare, Dovete semplicemente distogliere l'attenzione. Lo dovete trasformare in un emendamento, impedendo a un ramo del Parlamento di potersi esprimere, sperando in questo modo che tutto vada in dissolvenza. Questo è tipico degli ignavi.

non si è detto che vi volevate nascondere, che volevate fuggire, che eravate ignavi; per non parlare di paragone di carattere zoologico. Ringrazio il senatore Lombardo per la sua preziosa lezione. Visto che è così efficace, io lo invito a fare le stesse lezioni in Svezia, dove hanno espulso persone verso l'Iraq; o in Germania, dove li hanno mandati in Afghanistan, un Paese sicurissimo, governato con grande equilibrio dai talebani; o in Olanda, dove hanno espulso persone verso la Siria. Visto che queste cose sono così palesi, le vada a spiegare: a meno che, nella sua sapienza, lei sappia che Svezia, Germania ed Olanda sono uscite dall'Unione europea. Infine, come ha detto qualcuno assai più bravo con l'italiano di me, il "sugo" della storia è che in quest'Aula c'è una parte politica che non vuole che, in nessun modo, nessuno mai degli immigrati, qualunque sia la situazione, possa essere espulso. Di conseguenza, forse i loro elettori ne prenderanno atto.

sull'andamento dei lavori in Commissione, che peraltro avevano visto anche una prima anticipazione nella Conferenza dei Capigruppo, trovando comunque attenzione e sensibilità. Evidentemente,

per chi l'ha sostenuta - solo per riportare correttamente - di democrazia sostanziale. Questa verrà riportata, come è stato chiesto, alla Presidenza, esattamente nei termini usati da tutti coloro i quali sono intervenuti in quest'Aula.

la fissazione di obiettivi chiari su dove si deve andare. Infatti, caro Ministro, modificare in meglio le norme va bene, ma bisogna far capire dove un provvedimento di questo tipo vuole portare, al di là del fatto che era ora di fare una norma che riguardasse la montagna, ma se non si capisce dove si va, anche questa norma è destinata a non avere grande successo. In tal senso propongo in questo emendamento di fissare un punto chiaro: il territorio montano, territorio delicato, è sì uno scrigno di natura ma, come ho provato a dire in un mio intervento precedente, rende necessaria la presenza umana

in equilibrio con le attività umane consentite. La natura non va conservata in quanto tale e basta, ma va conservata in modo tale che l'uomo che vive in montagna possa sviluppare un'esistenza dignitosa e di comunità. Ecco, questo è un passaggio che manca in questo provato a proporre con questo emendamento. Inoltre propongo un altro passaggio importante, a mio avviso. Per quanto riguarda i grandi predatori, questa norma non fa un granché. C'è un passaggio che, secondo me, va perlomeno meditato: il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, nel 2017 fece un'ordinanza per abbattere un orso con un'istruttoria lunga decine di pagine e venne denunciato e rinviato a giudizio dal tribunale penale perché, secondo la procura e secondo chi lo accusava, contravveniva

Ora mi domando: se un Presidente fa fare un'istruttoria e presenta un atto con una serie di allegati che motivano le ragioni per cui quell'atto è stato firmato, come si può ipotizzare, anche solo per buonsenso,

di ovviare a siffatta possibilità: non che l'atto non possa essere illegittimo, ma sarà illegittimo dal punto di vista amministrativo. Che configuri un reato è veramente una cosa che può succedere solo nel nostro Paese. Il mio emendamento ha questo fine.

"Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «All'interno di un quadro di conservazione nazionale ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è definito annualmente, su base regionale o delle province autonome, il tasso massimo di prelievi tale da non pregiudicare il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie Canis lupus cui fare riferimento ai fini delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della Direttiva 92/43/CEE. Il decreto di cui al periodo precedente è emanato entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.»".

intervengo per sottolineare, riprendendo quanto oggi ha detto il senatore Borghi

a proposito dell'istituzione di un tavolo tecnico al quale dovrebbero sedere il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, il Commissario per il contrasto alla siccità e e i Presidenti delle Regioni invitati. Qui si pone di nuovo il tema dell'articolo 81 come un'idea di costi incrementali per aiutare i Ministri e i Presidenti delle Regioni a fare il proprio dovere d'ufficio, cioè a riunirsi per analizzare un problema. Vorrei precisare che, quando noi parliamo di tavolo tecnico, intendiamo una riunione tra persone che devono lavorare; non c'è un acquisto di mezzi mobili e, quindi, del tavolo medesimo o delle sedie. Battute a parte, questo dà un'idea. Questi emendamenti noi li abbiamo presentati per dimostrare l'assenza di analisi e di disponibilità al dialogo della maggioranza con l'opposizione. Di fronte a emendamenti di questo tipo,

è già in essere; non c'è bisogno dell'emendamento perché si sta già affrontando la questione; oppure dovreste dire certamente sì, perché è una volontà del Governo affrontare queste emergenze al più presto possibile e, quindi, volete dare un segnale politico approvando un emendamento che è a costo zero. Rifugiarsi invece nell'articolo 81 per respingere la costituzione di un tavolo tecnico che politicamente significa banalmente riconoscere l'emergenza della siccità nel Sud e nelle isole significa ancora una volta confessare l'inerzia politica, l'incapacità di ascoltare i bisogni del Paese e di confrontarsi costruttivamente con le minoranze. È la confessione dell'inattività di questo Governo e - non voglio nemmeno dirlo - della mancata lettura dei nostri emendamenti.

intervengo sull'ordine dei lavori. Credo che a questo punto ci sia un problema procedurale piuttosto serio, la relatrice ha comunicato all'Assemblea che sugli emendamenti 16.0.150 e 16.0.151 1.12 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81

sono emendamenti procedurali, che non hanno alcun onere, di alcuna natura. Mi chiedo a quale titolo si apponga l'articolo 81 su interventi procedurali. Uno è una delega al Governo, che peraltro ripropone una delega già in passato trasformata in legge e poi lasciata decadere. Quindi, si sarebbe dovuta dichiarare *ab origine.* Un'altra è un'attività connessa con l'impiego di risorse già esistenti.

Commissione, legittimamente. Su di esso, però, la Presidenza nulla può eccepire, se non prendere atto sia del parere della 5a Commissione che delle sue obiezioni. Quindi, da questo punto di vista, non possiamo che procedere oltre. Spero di essere stata esaustiva, anche se non soddisfacente

Presidente, al di là della *querelle* che abbiamo avuto

il testo di una legge della Regione Piemonte, approvata da una Giunta di centrodestra un po' di anni fa. Si tratta di una norma che - a mio giudizio - ha funzionato e, anche per evitare di cadere nel balletto delle posizioni, penso che, quando si fanno delle norme che funzionano, bisogna avere il il coraggio di dire che debbono essere riproposte. Mi sorprende che qui il centrodestra voti contro una disposizione che ha approvato altrove.

Dire che almeno il 3 per cento di quei proventi debbano essere destinati ad attività di tutela dell'assetto idrogeologico sembrerebbe una cosa scontata. previsioni andrebbero a tutela delle sorgenti, delle opere di captazione, del drenaggio delle acque e della riproducibilità del bene. Francamente non si capisce il motivo, se non un'ostilità preconcetta nei confronti della minoranza che ha proposto questa soluzione, per il quale si vuole votare contro. È di tutta evidenza che, se noi non introduciamo, in una logica di finanziamento ordinario e costante, il meccanismo della tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano, e ogni volta ci affidiamo a provvedimenti straordinari affidati alla finanza pubblica - che una volta ci sono, una volta non ci sono, una volta arrivano, una volta non arrivano - non riusciremo a portare a sintesi un tema di così grande valenza; tema che, peraltro, segnalo verrebbe sviluppato dai Comuni, dalle Unioni dei Comuni e dalle Comunità montane assicurando anche un ritorno economico, sui territori, dalle opere di manutenzione. Mi sembra che sarebbe una misura di buonsenso e non riesco a comprendere il motivo per il quale, pervicacemente, ci si ostina a dire di no.

Signora Presidente, dal punto di vista procedurale qui siamo di fronte a qualcosa di piuttosto curioso. In genere il Governo chiede poteri al Parlamento Parlamento e alla propria maggioranza. Noi invece ci troviamo in una condizione nella quale è la minoranza a chiedere al Governo di fare qualcosa in termini di poteri e il Governo dice no. Sia chiaro che io non voglio fare questa cosa qui: siamo veramente in un'operazione di rovesciamento dei fattori. Allora è piuttosto curioso e singolare che il Governo si rifiuti di dar corso - e qui vengo al merito della questione ad una procedura di introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali, che è una misura già in corso in diversi Paesi avanzati e che stabilisce sostanzialmente un principio semplice: nel momento in cui i territori producono, attraverso un'azione di natura ecosistemica, dei benefici dal punto di vista non solo naturalistico, ma anche economico, è giusto che una parte di questo ritorno economico possa ritornare ai territori per assicurare la tutela e la salvaguardia di questo bene. Cito il caso di scuola più clamoroso: il servizio ecosistemico che la città di New York paga alle contee che gli assicurano l'acqua ai fini idropotabili. Siccome la città di New York non ha in sé la capacità di drenare e di depurare tutto quel bisogno del fabbisogno che ha, è costretta a ricorrere a territori che producono questo bene. Quei territori non possono fare evidentemente un certo tipo di sviluppo, perché depaupererebbero e comprometterebbero la capacità di produrre quel tipo di bene comune. Quindi che cosa fa la città di New York? Paga Paga quei territori per rimanere così, per consentire la riproducibilità del bene. È un'operazione che non c'entra nulla con la finanza pubblica, perché è un accordo tra consumatori e produttori che consente un'operazione di tutela e di salvaguardia ambientale e di riproducibilità del medesimo. Siccome questi temi esistono e nei Paesi più avanzati (penso ad esempio alla Svizzera) da anni producono delle risposte, ci sembrava piuttosto naturale che il Governo potesse essere investito dello studio e della predisposizione di questo tipo di funzioni in maniera tale che i territori potessero beneficiare di queste rimesse. Invece, si preferisce stare dentro una dimensione da finanza derivata, forse perché in questo modo si controllano meglio le filiere di potere connesse al denaro pubblico. E anche qui torniamo indietro anziché andare avanti.

1. Al fine di incentivare l'insediamento di nuovi residenti nei piccoli comuni delle zone montane con popolazione non superiore a 5.000 abitanti soggetti ad un costante decremento demografico rilevato dall'Istat nel corso degli ultimi tre censimenti generali della popolazione, è istituito un Tavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni e dei rappresentanti delle imprese che erogano i servizi di energia elettrica, gas e acqua, finalizzata a definire le modalità di riduzione delle tariffe per l'erogazione di energia elettrica, gas e acqua, commisurate al nucleo familiare trasferito e al reddito familiare. Per la partecipazione al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».".

Presidente, colleghi, quasi ogni giorno ci troviamo di fronte ad un femminicidio. Sono tragici episodi, brutali, che insanguinano tutto il Paese. In ogni angolo si innalza un grido di dolore, che risuona nella nostra Nazione. L'immagine di Sara Centelleghe, tragicamente assassinata con 30 forbiciate, ci impone una riflessione urgente e profonda. Dal gennaio 2024 le statistiche fornite dal Ministero dell'interno parlano chiaro. Sono state assassinate oltre novanta donne da uomini che dicevano di amarle, vittime di una cultura che continua a perpetuare la disuguaglianza e la violenza di genere. Questi dati non sono solo numeri; sono vite spezzate, sogni infranti e famiglie distrutte. Dobbiamo chiederci come possiamo migliorare e garantire che queste tragedie non si ripetano. Onorevoli colleghi e colleghe, c'è una risposta e non è solo di carattere legislativo, ma soprattutto culturale. È nostro compito pertanto agire con urgenza, al fine di educare le nuove generazioni e dare loro gli strumenti del vivere civile. Il termine femminicidio descrive non solo l'omicidio di una donna, ma anche e soprattutto un atto che svela il profondo radicamento della misoginia nella nostra cultura e questa non è altro che la punta dell'*iceberg* di una profonda angoscia che alberga nella mente e nei cuori di alcuni maschi, nostri padri, nostri fratelli o nostri figli, che fuggono dalla loro esistenza e dal dolore che imprigiona la loro mente. Bisogna avere il coraggio di eliminare in un sol colpo la differenza di genere almeno dal punto di vista economico.

le nuove generazioni al rispetto e all'uguaglianza e promuovere una cultura di non violenza. Tutti hanno un ruolo cruciale in questo processo: le scuole, le famiglie e le istituzioni. Torno a proporre l'introduzione dell'educazione emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado. È auspicabile che la violenza e il femminicidio diventino solo un doloroso ricordo del passato, un vero tabù. Non c'è più tempo, bisogna investire nell'educazione emotiva per formare una nuova generazione consapevole e sensibile per coltivare una nuova dimensione di vita, al fine di affermare la convivialità. Ricordiamo i nomi delle ultime cinque donne assassinate, che potrebbero essere nostre mamme, nostre sorelle, nostre figlie: Sara, Aurora, Flavia, Marina e Celeste. Siano esse di monito per darci la forza e il coraggio di agire. Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo lavorare insieme, senza steccati politici, per costruire una società più giusta e sicura,